nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà. da tempo un convinto assertore del monocameralismo: una sola Camera politica che dà la fiducia al Governo, una Camera delle Regioni che entra nel processo legislativo come espressione dei legittimi interessi del sistema delle autonomie. Ma nel corso di questi lunghi e purtroppo, almeno sul punto, del tutto inconcludenti dibattiti sui vizi e i pregi dell'italico bicameralismo perfetto, mi sono spesso dovuto arrendere di fronte alla forza dell'unico argomento a mio giudizio valido, avanzato dai sostenitori del bicameralismo stesso: quando una Camera sbaglia, ad unanime giudizio, l'altra interviene e corregge, facendo in realtà risparmiare tempo e denaro alla Repubblica. Ora, signor rappresentante del Governo, colleghi della maggioranza, una cosa è certa: in questo decreto, alla Camera, avete infilato norme che non noi, ma voi considerate sbagliate, da espungere o da modificare. Ripeto: norme che voi considerate sbagliate e che infatti il Governo ha già deciso di eliminare o di cambiare, convinto dall'intervento equilibrante e di garanzia del Capo dello Stato, che voglio tornare a ringraziare, prendendo esplicitamente le distanze dalle critiche pretestuose e senza fondamento che l'Italia dei Valori ha voluto rivolgergli ancora in questa circostanza. Ma ecco il punto: il Governo - che deve cambiare queste norme e ha già deciso quali norme cambiare e perché cambiarle non consente al Senato della Repubblica né di fare la scelta più dignitosa e lineare, ossia di votare i tre o quattro emendamenti in questione chiudendo la conversione alla Camera entro lunedì prossimo, né di fare la scelta - poco dignitosa certo, di fare la scelta - poco dignitosa certo, ma almeno trasparente - di approvare in questa sede un atto di indirizzo al Governo che minuziosamente indichi le correzioni da apportare attraverso un nuovo decreto. Né l'una, né l'altra delle scelte. Il Governo ha scelto di intraprendere la strada - si potrebbe dire, parafrasando il titolo di un famoso libro di economia - della produzione di decreti attraverso decreti. Ieri, colleghi della maggioranza, durante la discussione nelle Commissioni bilancio e finanze riunite abbiamo fatto un ultimo tentativo di salvarvi la faccia, chiedendo al ministro Tremonti, che era presente alla nostra discussione, di dire al Senato quali correzioni il Governo avesse in animo di apportare al decreto. Ma il Ministro non ha risposto. Così, colleghi senatori della maggioranza, sarete vittime di un clamoroso paradosso: voi sarete, nella penosa cronaca di questa che è la più grande recessione del dopoguerra, come quelli che volevano approfittare della crisi per bloccare nove su dieci - così si legge sui giornali di questa mattina - delle indagini in corso presso la Corte dei conti contro amministratori pubblici infedeli o dolosamente incauti, mentre il Governo, in quella stessa cronaca, ci starà almeno formalmente come quello che ha impedito a voi, cioè ai senatori del PdL e della Lega, di colpire così duramente gli interessi della Nazione. Oppure, per fare un altro esempio, forse di più immediato effetto, voi, senatori del PdL e della Lega, starete nella cronaca di questa crisi come quelli che volevano approfittarne per imporre ai terremotati dell'Abruzzo di pagare tra cinque mesi il 100 per cento delle imposte sospese dopo il terremoto, mentre il Governo ci starà come quello che, alla fine, si sarà convinto che questa è pura follia e vi avrà messo in qualche modo rimedio. Verrebbe da dire: contenti voi! Forse però è più utile porci una domanda: cosa spiega il ricorso ad una scelta così umiliante per l'istituzione Senato e le persone stesse dei singoli senatori della maggioranza da parte del Governo? Ad essere sincero, non credo che il generale agosto vi entri granché. Anzi, la minaccia del generale agosto sarà più grave tra 15-20 giorni, quando si tratterà di convertire l'annunciato decreto "correggi disastri". Spiega molto di più secondo me, rispetto al generale agosto, la politica. Non so se sia già finita la luna di miele tra Governo e Paese. Purtroppo, per la verità, non lo credo. So per certo, però, che su due temi - politica estera e politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno - stiamo assistendo da settimane ad una seria incrinatura del rapporto tra Popolo della Libertà e Lega e ad un relativo, ma significativo indebolimento della *leadership* di Berlusconi. Ecco perché il Governo ha avuto paura di tornare alla Camera e forse ha addirittura paura di aprire a qualche modifica qui al Senato. I numeri delle recenti votazioni alla Camera giustificano questa paura. Ma sono i numeri sulla gestione del FAS. (Fondo per le aree sottoutilizzate), finalmente resi noti ieri dal Governo, anche grazie alla nostra insistenza nelle Commissioni 5a e 6a del Senato, a dare conto del fondamento delle contraddizioni che si stanno aprendo nella maggioranza. I numeri che citerò sono tutti relativi alla competenza giuridica, perché sulla cassa il Governo ha formalmente dichiarato di non poter dare informazioni al Parlamento. Torno così a dire che a mio giudizio, in questo momento (ecco cosa spiega tutto questo andirivieni di cifre inconcludenti che si pubblicano sui giornali in questi giorni) sotto il profilo della cassa, la gestione prevede 370 milioni di euro e non un euro in più. Quindi, siamo praticamente ad aver azzerato le disponibilità di cassa sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Comunque, parliamo della competenza giuridica.

qui il Governo svolge una funzione di mero coordinamento, ma questi sono soldi delle Regioni, dei programmi regionali. Qui il Governo non concede nulla, signor Sottosegretario, non toglie nulla per la banale ragione che non può né concedere né togliere, perché non sono soldi suoi. Può - e deve, a mio giudizio - svolgere rispetto al passato (ciò vale per tutti i Governi, e non solo per questo ovviamente) una più forte azione di coordinamento, di concentrazione degli obiettivi, di coordinamento interregionale. Ma sono soldi delle Regioni. Per i programmi gestiti dalle amministrazioni centrali il FAS prevede (competenza giuridica) 25,4 miliardi Qui, sì, decide il Governo, con un vincolo di legge: l'85 per cento deve essere allocato al Sud. Non perché lo dice il senatore Morando, ma perché lo dice la legge.

Fondo infrastrutture, 12,3 miliardi; Fondo per gli ammortizzatori sociali (Fondo sociale), 4 miliardi; Fondo strategico per l'economia reale, 9 miliardi. Del Fondo strategico, 4 dei 9 miliardi sono stati allocati per finanziare l'intervento sul terremoto in Abruzzo. Lo sottolineo per dire che, per la prima volta nella storia delle calamità naturali di questo Paese, la solidarietà del Paese a favore dei terremotati è interamente a carico delle popolazioni del Mezzogiorno. Forse bisognerebbe almeno dire loro grazie! Forse almeno un grazie glielo dovremmo a quelle popolazioni, che sono quelle che stanno peggio in Italia ed alle quali abbiamo messo a carico integralmente la solidarietà nazionale per l'intervento post‑terremoto. 4 miliardi per l'Abruzzo. Il resto, tra decreti e delibere del CIPE, è stato allocato in modo tale che restano da allocare 2 miliardi di euro. Ripeto, sto leggendo la Nota del Governo: si di 2,1 miliardi. Ho visto questi numeri e ho sentito che ieri il Presidente del Consiglio ha detto che il prossimo piano per il Sud sarà chiamato «piano Berlusconi». Lo annuncia «Il Messaggero» di oggi: «I miei vogliono sia intitolato a me», ha detto il Presidente del Consiglio.

il Fondo Matteoli è dotato di 12,3 miliardi di euro, il Fondo Letta di 9 miliardi di euro il Fondo Sacconi di 4 miliardi di euro, mentre il suo, il Fondo Berlusconi (nuovo conio), potrà essere dotato, al massimo, di 2 miliardi. Non vorrei essere nei panni di colui che nelle prossime ore dovrà andarglielo a dire. dire. Questa è la realtà dei fatti: altro che "Ora i soldi e i piani per il Sud"! Lo dice il Governo, non il senatore Morando: ora i soldi per il Sud sul FAS non ci sono più, perché sono stati spesi per fare altro. Il problema è che chi è stato zitto ed ha avallato le scelte che hanno condotto a questo esito potrà oggi meritarsi forse qualche titolo di giornale del chiacchiericcio politichese che caratterizza il confronto politico in Italia, ma non avrà modo di recuperare il danno che ha contribuito a provocare. Infine,

Sud. Mi chiedo, vi chiedo, e chiedo anche al Ministro dell'economia: ma si può costruire dal nulla una banca (approfitto di avere di fronte, come interlocutore, il senatore Dini, che certo di queste cose ne sa più di me),

Lasciamo perdere quindi la propaganda e proviamo a fare un discorso serio sul problema della Banca del Mezzogiorno. la sua banca ce l'ha già, ed è sua davvero, non deve essere creata: è un'azienda di credito inserita in uno dei più grandi gruppi bancari europei, cioè Intesa‑San Paolo. Quella banca si chiama Banco di Napoli. Ha ritrovato il suo nome, la sua originaria ragione sociale, ma ora, nel rispetto dell'appartenenza ad un grande gruppo nazionale, deve davvero diventare la banca regionale del Mezzogiorno continentale. Una vera banca capace di agire nel *retail*, nel corpo rete e nella gestione del sistema dei pagamenti. Il Banco di Napoli non è, e non può restare semplicemente, una delle 22 banche locali della rete di questo grande gruppo, il principale italiano. Il socio di controllo del Banco dovrebbe dunque aprire il capitale agli attori economici locali, favorendo la diffusione dell'azionariato tra famiglie e imprese, riportando in prospettiva in Borsa il titolo del Banco. La stessa Fondazione Banco di Napoli dovrebbe rientrare nel novero degli azionisti, indicando, anche simbolicamente, che è finita una stagione di penalizzazione delle realtà locali e ricostruendo un legame oggettivo con un passato che, a questo proposito, affonda le proprie radici nella stagione dei governi del Mezzogiorno degli Aragona, nel secolo XV. Il Governo deve dunque smettere con la propaganda facile e utilizzare, anche a questo proposito, la forza di persuasione, non solo morale, che oggi ha nei confronti del sistema delle banche, e certamente anche nei confronti del Gruppo Intesa, per agire in questa direzione. Sarà un modo per tentare di passare, dopo un anno di facile propaganda, ad affrontare i problemi, che sono difficili, che questo Governo ha semplicemente rinviato nel tempo venendo in questa sede a chiederci la fiducia,

Presidente, onorevole Sottosegretario, siamo oggi qui a discutere della fiducia al Governo. Ieri discutevamo del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e della sua conversione in legge. Signor Sottosegretario, lei lo ricorderà, visto

blindato, impedendo al Parlamento di poter cooperare, maggioranza e opposizione insieme, per la costruzione di una buona legge, visto che di fatto stiamo parlando di una legge finanziaria. Stiamo parlando della vostra politica economica, che definirei un po' spezzettata, perché, come lei ci potrà confermare, illustre rappresentante del Governo, state facendo una politica economica articolata in vari provvedimenti - sette per la precisione, di cui quattro li avete definiti anticrisi - negli ultimi otto mesi.

martedì, il provvedimento licenziato dalla Camera a oggi, che è venerdì, avendo già esaurito il dibattito in Commissione, il voto sugli emendamenti e ora siamo sulla fiducia, e non più sul testo del decreto-legge n. 78. Perché Perché vi trovate in una condizione difficile, che è quella di chi, non sapendo più dove trovare i numeri esatti per le promesse che ha fatto ai cittadini italiani provare in un qualche modo a mantenerle, comincia a salire, ad arrampicarsi sugli specchi, quando invece avete una strada facile da seguire. Devo dire che in ciò vi abbiamo aiutato, perché più di un mese fa abbiamo licenziato in quest'Aula

Voi, invece di andare alla Camera e accelerare la trasformazione in legge di quel disegno di legge licenziato in questa sede in modo ampiamente *bipartisan* da maggioranza e opposizione, lo avete bloccato alla Camera. Perché lo avete fatto? Perché, invece di stare qua a discutere l'ultimo DPEF, ci metterete in condizione di non discutere il prossimo Documento di finanza pubblica (come si chiama nel nuovo testo

interne, e cioè quella famosa necessità di trasparenza dei conti pubblici che per 21 mesi vi abbiamo sentito criticare, dicendo che in realtà noi avevamo molti più soldi da parte che non volevamo

dei conti, un luogo tecnico e tecnologico dove gli Uffici studi di Camera e Senato, insieme alla Ragioneria, potevano far diventare questo Paese il fiore all'occhiello delle riforme e della capacità del Parlamento di interloquire da una posizione di pari conoscenza con il Governo. Quella mediazione voi l'avete bloccata per un problema di trasparenza dei conti, mantenendo tutti i numeri in possesso della Ragioneria e non mettendoli a disposizione del Parlamento. Ora ci troviamo a svolgere un dibattito sulla questione di fiducia perché questo decreto era blindato tre giorni fa ed è più blindato oggi. Ieri ci avete in qualche modo fatto capire

Se il problema è questo, allora ditelo che non riuscite più a tenere la maggioranza perché le vacanze sono più importanti della manovra finanziaria; avremmo così finalmente qualche dubbio che la vostra granitica schiera potrebbe in qualche modo bloccarsi. Vi è di più. Nel corso del dibattito di ieri si presenta improvvisamente l'uomo forse più autorevole di questo Governo dopo il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'economia e delle finanze. Immaginavamo venisse a dirci Immaginavamo venisse a dirci qualcosa in ordine ad un provvedimento normativo, cioè a un nuovo decreto-legge che dovrebbe modificare parti del decreto-legge al nostro esame (non mi soffermo su questo, perché potrei perdere minuti preziosi; del resto, lo ha già fatto molto meglio di me il senatore Morando). Invece no, questo Ministro, da tutti chiamato genio (ed effettivamente è una mente molto lungimirante) viene a dirci tre cose. La prima: scopriamo da ieri, signor Sottosegretario, che l'oro della Banca d'Italia non è più della Banca d'Italia, ma è degli italiani.

Mai avevamo sentito in un'Aula parlamentare di questo Stato democratico una baggianata simile. Invece l'avevamo sentita in un altro Stato: si chiama Argentina, un certo Paese dell'America Latina dove, in assenza dello Stato di diritto, si susseguono populisti che generano Governi di transizione e che mandano in *default* le casse dello Stato, oltre ai risparmi dei cittadini. Speriamo che questa non sia un'anticipazione di quello che è già accaduto in Argentina. La seconda cosa che ci dice il Ministro dell'economia e delle finanze

che sulle altre questioni non c'è nulla da dire. Allora chiediamo: che cosa è venuto a fare ieri il Ministro dell'economia e delle finanze? Eppure, entrava per la seconda volta in quest'Aula per dire qualcosa di importante. È venuto a dirci che l'oro della Banca d'Italia, non è della Banca d'Italia, ma è degli italiani? Ha fatto un'ulteriore operazione nei confronti della Lega? Ha fatto un'operazione di raccordo e di chiarezza? Che cosa ha voluto fare con quel passaggio? Vede, signor Sottosegretario,

caso. Siamo arrivati ieri sera finalmente a votare gli emendamenti nelle Commissioni riunite, non senza qualche difficoltà da parte vostra: i due relatori non erano presenti, abbiamo dovuto aspettare un bel po' prima che arrivassero, addirittura uno si è presentato - lo dico bonariamente, ovviamente dicendo che non era stato avvisato. Eppure noi eravamo qui in massa, fermi ad aspettare che voi raggiungeste il vostro numero per poter cominciare a votare. Grazie all'insipienza di alcuni colleghi di questa opposizione, non vi abbiamo mandato sotto nelle prime tre votazioni, visto che mancavano uno dei nostri senatori e due di un altro Gruppo dell'opposizione.

Voi non spiegate mai i problemi che vi poniamo, non vi impegnate nemmeno a dire che sono baggianate. Voi cambiate completamente argomento e tendenzialmente non rispondete oppure letteralmente parlate di altro (si parla di alfa e voi parlate di omega). È diventata una vostra abitudine quella di comunicare al Paese le non risposte a chi prova umilmente a fare il proprio dovere in queste Aule del Parlamento per poter trasferire ai cittadini un minimo delle cose importanti che si vogliono fare nell'interesse pubblico. Voi invece non rispondete mai.

genericamente identificate in circa 3-3,5 miliardi di euro dovrebbero servire per la manovra. Avete innovato in materia di giudizio di responsabilità sulla Corte dei conti. Ieri vi abbiamo posto dei problemi nei luoghi in cui si esaminano pacatamente le questioni - come ci dite voi

fanno. Per l'Italia, a parte la Regione Abruzzo e qualche soggetto che se ne interessa, il terremoto non c'è più, perché voi continuate a parlare di cose positive e risolte. Avete aperto un budello di strada per tre ore e avete detto di aver riaperto il centro storico, mentre dentro c'è il vuoto cosmico. Anzi, può chiedere cortesemente al ministro

Dove sono le forze dell'ordine? Mi risulta che a settembre verranno via tutte le forze aggiunte dal mese di aprile: perché, è cambiato qualcosa? Abbiamo ridato vita a quella città? Niente. Su questo e su altro, signor Sottosegretario, voi non rispondete. Non rispondete sulla questione delle imposte. Lei sa personalmente quanto io la stimi,

tutte le cose che voi avete erroneamente scritto in merito alla restituzione delle imposte, per i motivi che ormai sappiamo. Avete chiesto agli abruzzesi una restituzione del 100 per cento

che oggi state convertendo? Avete rivoluzionato anche le fonti di diritto? Ciò nonostante, le immagini della televisione non danno la possibilità di spiegare tutto questo, ma fanno vedere che ieri il presidente del Consiglio Berlusconi ha messo una bandiera

compresa L'Aquila) non state realizzando niente? Perché non rispondete ai Sindaci che vi riconsegnano la fascia - e non sto parlando di Cialente, ma dei Sindaci dei piccoli centri centri - e non realizzate nulla di quello che sbandierate e che dite di aver fatto? Perché non parlate della droga nei campi e delle scuole che non riaprite? Avete aperto una tenda un mese dopo il terremoto e avete detto che avevate aperto tutte le scuole. Perché non dite che la gente non rientra nel proprio Comune perché deve iscrivere i figli nella scuola sulla costa e per farlo deve lavorare deve lavorare lì, deve stare vicino ai propri figli e non rientrerà più dentro L'Aquila? Perché non spiegate queste cose? Perché non modificate in questo decreto-legge, o nel prossimo che correggerà questo, le cose che avete sbagliato?

Ma arriverà un giorno, come per tutti, signor Sottosegretario, com'è arrivato per noi e per la nostra maggioranza, che è crollata sotto inutili litigi andati avanti per 21 mesi, in cui anche le vostre mancate verità verranno alla luce e sarà un giorno di chiarezza per tutti.

secondo i dati ISTAT), il Governo ha partorito un decreto anticrisi - sul quale, mortificando la funzione parlamentare, ha chiesto il ventitreesimo voto di fiducia - che non affronta i nodi reali del Paese, ma continua a strizzare l'occhio ai suoi sodali, quali banchieri, assicuratori, Confindustria, monopolisti elettrici e del gas, cartelli organizzati, evasori, riciclatori e faccendieri, con i quali continua ad andare a braccetto. Mentre secondo tutti gli indicatori economici l'uscita dalla crisi non sarà breve né indolore, il Governo continua a professare ottimismo di facciata, sperando che «passi la nottata», appioppando patenti di catastrofismo a tutti coloro che osano dissentire. Non ci sono solo i dati OCSE a confermare l'irrilevanza delle misure stanziate in funzione anticrisi, pari a percentuali microscopiche del PIL, ossia 85 milioni di euro nel 2009, 2.102 milioni nel 2010 contro una media del 3,9 per cento del PIL dell'area OCSE. Ci sono anche altri dati che misurano la profondità della crisi, come le sofferenze bancarie, che hanno raggiunto il record di 46.398 milioni di euro ad aprile (1.631 in più di marzo 2009), con un rapporto tra sofferenze nette e patrimonio di vigilanza pari ad oltre il 9 per cento, quasi un punto in più sul 2008. C'è ancora incertezza sull'impatto della recessione e sulle sofferenze, come ha detto Bini Smaghi, membro della BCE. Il sistema bancario - ha aggiunto - non riesce ancora a finanziarsi a medio lungo termine, perché la fiducia del mercato non è stata ristabilita. Il rischio è che quando l'economia si stabilizzerà e mostrerà segni di ripresa, il sistema bancario non sia pronto a sostenerla, perché se non riescono a trasferire l'ingente liquidità al sistema delle imprese, significa che la loro posizione patrimoniale non è a posto: queste sono Per non parlare dei crediti incagliati che, seppur non rilevati statisticamente, possono ammontare a 100 miliardi di euro. Per non parlare delle cartolarizzazioni: nel 2008 gli attivi ceduti dai principali gruppi bancari italiani nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sono triplicati, da 40 a 120 miliardi di euro. Queste operazioni hanno avuto ad oggetto in prevalenza mutui e crediti commerciali. A questa attività si somma quella realizzata attraverso le prime operazioni di emissione di *covered* *bond* da parte di banche italiane per un ammontare complessivo di 6 miliardi di euro. Insomma, la crescita delle cartolarizzazioni ha determinato un aumento delle esposizioni da 70 a 130 miliardi - mentre le operazioni di dubbia esigibilità, impacchettate quasi come i *subprime* e date in garanzia alla BCE a fronte della concessione di liquidità, continuano ad aumentare. anticrisi vi sono pochissime misure condivisibili, come la penale sui mutui, nel caso in cui la surroga non si perfezioni, o come i tempi certi per ricevere bonifici e assegni circolari. È infatti un decreto contraddittorio, che fa finta di combattere l'evasione con la possibilità di accedere a dati e informazioni della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'ISVAP, ma subito introduce lo scudo fiscale e la tassa sull'oro, prevedendo che le plusvalenze derivanti dall'oro e da altri metalli siano tassate al 6 Non era meglio dismettere oro e riserve della Banca d'Italia, così come hanno fatto tutti gli altri Paesi dell'eurosistema da tempo, appostando il ricavato alla riduzione del debito pubblico?

anche sugli sconfinamenti. Un'altra questione riguarda la svalutazione dei crediti in sofferenza, un altro regalo alle banche, che sale infatti dallo 0,30 allo 0,50 per cento. Inoltre, viene ridotto da 18 a 9 anni il periodo in cui è ripartita la deduzione della quota che supera tale tetto. Meno male che il Ministro dell'economia sostenne qualche mese fa, in Commissione finanze, proprio qui al Senato, che «I banchieri che sbagliano o vanno in galera o vanno a casa». I banchieri, a distanza di mesi, ancora tutti in carica ed a piede libero, continueranno a percepire il "pizzo" sulla commissione di massimo scoperto.

indicatore, il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che avrebbe imposto alle banche trasparenza informativa a favore delle piccole e medie imprese e dei cittadini ed effettiva concorrenza tra gli istituti di credito. Il cittadino o il piccolo imprenditore che si fossero presentati in banca per chiedere un prestito avrebbero ricevuto il tasso reale applicato, comprensivo di qualunque tipo di costo, spesa o commissione. Sarebbe stato uno strumento innovativo e rivoluzionario, ma questa cosa cosa è stata cancellata la mattina dopo. Inaccettabile lo slittamento di un anno, ossia fino al 1° gennaio 2011, del divieto di commercializzare i sacchetti di plastica. Vergognoso - e lo abbiamo detto - il lodo Bernardo,

segnalato anche dalle procure regionali della Corte dei conti che esercitano l'azione per il risarcimento del danno, è scritto è scritto che la Corte potrà perseguire il danno erariale «di uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione», il che significa restringere l'area dei soggetti indagabili e tirar via d'un colpo municipalizzate, enti mutualistici, comunità montane, e perfino la Banca d'Italia. Come ogni buona legge *ad personam*, anche il lodo Bernardo si applica ai processi in corso. Incomprensibile l'articolo 17, comma 2, che autorizza Lazio, Campania, Sicilia e Molise a ristrutturare le operazioni in derivati, quello stesso Ministro che, dopo averli autorizzati nella finanziaria del 2001, ha definito questi strumenti la peste del XXI secolo. Dopo aver accertato che gli enti locali sono stati frodati e soffocati da 35 miliardi di debiti in derivati dove è il banco che vince sempre - dopo le inchieste di decine di procure e la chiusura delle indagini da parte del pubblico pubblico ministero Alfredo Robledo che indaga sulla ristrutturazione dei debiti del Comune di Milano, dove alcune primarie banche hanno lucrato ulteriori 100 milioni di euro addossati alla collettività con manager che, dopo aver guadagnato 3,4 milioni di euro l'anno secondo sistemi incentivanti fraudolenti, ne facevano vanto, come risulta dalle intercettazioni depositate, addirittura dandosi appuntamento a cena per festeggiare a *champagne*,

Lo scudo fiscale, come hanno scritto giornalisti attenti e con la schiena dritta, sarà l'apoteosi di furbetti e furboni di ogni categoria: migliaia di evasori grandi e piccoli, gli stessi che hanno nascosto oltre frontiera il tesoro di famiglia, si preparano a cavalcare il condono gentilmente concesso dal Governo Berlusconi. Prima hanno evaso il fisco adesso sono pronti ancora a truffare lo Stato. In altre parole, imprenditori, professionisti, finanzieri e manager faranno la cresta sui soldi che tornano in patria, sfruttando le norme che regolano il rimpatrio del denaro nero.

avvocati d'affari, fiduciari svizzeri e vari faccendieri, che da tempo si stanno attrezzando per far fronte alle richieste dei loro clienti. Proliferano i giochi di sponda estero su estero, alimentati con i prestiti di banche compiacenti, e le valutazioni gonfiate dei beni patrimoniali (case, gioielli ed opere d'arte): insomma, è come dire che lo Stato rinuncia ad ogni pretesa su quei soldi; si tratta di un vero condono tombale, un'offerta che non si può rifiutare.

Se l'evasore dovesse possedere fondi neri in Italia, ma non avesse ancora trovato il tempo e il modo di trasferirli all'estero, può farsi prestare i soldi su un conto estero per un importo pari a quello nascosto in Italia e poi riportare il tesoretto in Italia sfruttando lo scudo, senza svelare all'erario il reale ammontare del capitale rimpatriato. I margini di manovra sono ancora maggiori quando l'operazione di rientro riguarda attività non finanziarie (come case e, soprattutto, gioielli ed opere d'arte). Voglio ricordare che altri Paesi

del frutto di proventi che non si sa da quale destinazione vengano. Questo è uno schiaffo anche alla povera gente, alle piccole botteghe artigiane o a quei baristi che aprono i loro locali la mattina presto: diciamo sempre che bisogna fare la lotta all'evasione fiscale e rilasciare le ricevute fiscali, ma qualora essi non dovessero rilasciare uno scontrino per pochi euro si vedono chiudere i loro esercizi commerciali. Questo è il Governo, signor sottosegretario Giorgetti: ci complimentiamo con voi, signori della maggioranza e del Governo, per il vero capolavoro del decreto anticrisi; scudate e riciclate i capitali come ulteriore forma di condono tombale, facendo pagare una penale del 5 per cento - al contrario dei BOT, dei BTP e dei CCT, che pagano una ritenuta del 12,5 spremendo, al contrario, i contribuenti onesti, ai quali addossate un insostenibile peso fiscale, pari al 43,4 per cento, tra i più alti dei Paesi OCSE.

e neanche quei Ministri che voi avete giudicato dei vampiri hanno portato la pressione fiscale ad un livello così elevato. Mettete la mordacchia alla Corte dei conti che non potrà più indagare per danno erariale; regalate i soldi ed una scialuppa di salvataggio ai banchieri amici, con i quali continuate ad andare a braccetto e che potranno continuare indisturbati a frodare i risparmiatori ed a strozzare la clientela e le piccole e medie imprese, elargendo al contrario fior di finanziamenti dopo l'abusiva concessione del credito allegramente effettuata da banchieri, che sono diventati vostri amici, quali i Passera e i Profumo, ad amici e sodali come Zaleski e Zunino. Chiedete alle popolazioni abruzzesi con abitazioni e redditi distrutti dal terremoto di pagare tasse ed arretrati a partire dal 1° gennaio 2010, e non esiste ordinanza di protezione civile che possa rassicurarci.

di una manovra economica e di un decreto-legge anticrisi che, come al solito ispirati ad un Robin Hood alla rovescia, o meglio al Principe di Valacchia, finiscono per avvantaggiare i ricchi continuando ad impoverire i lavoratori, le famiglie, le piccole e medie imprese, la povera gente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è ormai da molto tempo che il mondo dell'economia e della finanza, unito alle organizzazioni sindacali, denuncia il grave stato in cui si trovano le imprese italiane. Anche il governatore

Un'attenta e obiettiva osservazione della vita economica e sociale del Paese ci fa capire quanto profondo è il malessere. Quindi, bisogna mettere in atto azioni efficaci ed efficienti. Ricordo che l'ANCI, consapevole della gravità della situazione generale nella quale versano i Comuni e a garanzia delle popolazioni amministrate, aveva rivolto un appello al Governo con il quale chiedeva una serie di interventi urgenti per consentire, in deroga al Patto di stabilità interno, l'utilizzo immediato dei residui passivi per la spesa in conto capitale, l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale, l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio per finanziare la spesa per investimenti la garanzia per la stabilità delle entrate comunali attraverso la compensazione dei tagli ai trasferimenti e la mancata integrale copertura degli interventi sull'ICI. Il Partito Democratico, con una mozione

per finanziare opere già progettate, cantierabili o già cantierate ma ferme a causa dei vincoli posti dal Patto di stabilità, e di adottare provvedimenti legislativi urgenti per garantire le immediate modifiche delle norme attuali che regolano i vincoli. Inoltre, abbiamo chiesto di creare una corsia preferenziale per l'utilizzo dei fondi residui passivi per la spesa in conto capitale, già a disposizione degli enti, da impegnare nella manutenzione dei luoghi pubblici (scuole, reti idriche, edilizia residenziale

con la speranza che la maggioranza ed il Governo vogliano predisporsi all'ascolto e al confronto costruttivo in un momento in cui il Paese chiede coesione sui temi economici senza barriere ideologiche. purtroppo prendere atto che, nonostante i numerosi appelli e le tante iniziative parlamentari promosse dal Partito Democratico, il Governo si è sempre rifiutato di prestare ascolto, intraprendendo iniziative legislative che delegittimano il Parlamento nelle sue funzioni, facendo quasi sempre ricorso a modalità poco ortodosse - oggi è l'ennesima riprova

Voglio ancora ricordare che al fine di scongiurare il collasso delle piccole e medie imprese è stato presentato ed accolto in quest'Aula, a luglio dello scorso anno - dunque non soltanto il ministro Tremonti riesce a guardare oltre l'economia

Ci rendiamo conto che parliamo di una somma tra i 40 e i 50 miliardi di euro non pagati alle piccole e medie imprese? È paradossale: sono le piccole e medie imprese che oggi finanziano lo Stato italiano perché, se quei soldi fossero nelle casse delle imprese, vorrebbe dire che queste potrebbero non rivolgersi alla banche e che, invece, lo Stato avrebbe necessità di pagare: e pagare vuol dire fare cassa. Invece, le imprese sono costrette a rivolgersi al sistema bancario.

misura del 3 per cento per aumenti di capitale che viene detassato per un importo fino a 500.000 euro. Allora, voi vi rendete conto che un imprenditore

*(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, noi ci troviamo, per l'ennesima volta, di fronte a un utilizzo anticostituzionale del Parlamento da parte di questo Governo. Vi ricordo, per l'ennesima volta, che l'articolo 81 della Costituzione attribuisce al Parlamento la funzione di indirizzo e di controllo in merito alla destinazione ed allocazione delle risorse pubbliche. Invece, il Governo qui comanda e questa maggioranza ratifica acriticamente. Voi state approvando a colpi di fiducia un provvedimento che sapete già verrà modificato con un decreto correttivo, sconosciuto ai più, che modificherà questo testo. Avete esautorato il Parlamento e lo avete svuotato delle sue prerogative. State facendo carta straccia della nostra Costituzione ma, quel che è peggio, in questo momento di difficoltà state tradendo i cittadini italiani. I dati presentati ieri dall'ISTAT descrivono un'Italia molto lontana dalle affermazioni ottimistiche del Presidente del Consiglio e di questo Governo. Quei dati dicono che l'occupazione nelle grandi imprese a maggio ha registrato un calo dello 0,3 per cento al netto della cassa integrazione guadagni, un meno 0,2 l'utilizzo della cassa integrazione ha visto un aumento del 10,8 per cento e che, rispetto a maggio 2008, è cresciuto di ben nove punti percentuali.

Il fenomeno è maggiormente diffuso al Sud, con una percentuale pari al 23,8 per cento, dove l'incidenza di povertà relativa è quasi cinque volte superiore a quella del resto del Paese, soprattutto nelle famiglie con due o più figli. Ma in questo provvedimento, purtroppo, non vi è traccia di risposte al Paese reale. C'è un'assenza totale di misure determinanti per lo sviluppo e la crescita. Il fatto più grave è certamente l'assenza di una politica di sostegno alla piccola e media impresa, al reddito dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie meno abbienti, indispensabile sia per il rilancio della domanda interna e dei consumi, sia per ragioni di equità sociale. Molte sono le criticità, tante le norme che andrebbero discusse e modificate. Avremmo dovuto, per il bene del Paese, trovare delle soluzioni comuni, invece oggi ci ritroviamo - così come è accaduto in questi giorni in Commissione lavoro per il parere - a discutere con una maggioranza sorda a qualsiasi richiamo. Tutto è già stato deciso altrove; sappiamo che questo provvedimento sarà modificato per esigenze di equilibri di Governo, prima con un maxiemendamento, su cui verrà apposta l'ennesima fiducia, e poi con un decreto correttivo, il tutto in tempi subordinati ad esigenze di chiusura estiva. L'Italia dei Valori aveva presentato in Commissione emendamenti migliorativi dell'articolo 1, proprio per dare maggior sostegno ai lavoratori in difficoltà. Avevamo proposto, per favorire i contratti di solidarietà, che la retribuzione del lavoratore al quale viene ridotto l'orario di lavoro

recuperando come copertura le somme dichiarate e non versate dai cittadini che hanno aderito alle sanatorie fiscali. Avevamo proposto di implementare l'istituto sperimentale di tutela del reddito, la prima forma di ammortizzatori sociali previsti per i collaboratori a progetto Co.co.co, istituita con il decreto-legge n. 185 del 2008, prevedendo una revisione delle condizioni per accedere a tale beneficio ed un'estensione a tutte le forme di lavoro atipico, nonché un incremento dell'indennità dal 10 al 30 Al contrario, il Governo non solo mantiene tutte le farraginose condizioni e i limiti per l'ottenimento dell'indennità, ma quel che è peggio, con il comma 8‑*ter* dell'articolo 1, finanzia ulteriormente il Fondo per l'occupazione e la formazione proprio con quei pochi fondi stanziati per l'istituto. La Banca d'Italia stima che i lavoratori dipendenti o parasubordinati che non hanno diritto ad alcun tipo di ammortizzatore sociale siano circa 1.600.000 e ci ricorda che nelle famiglie in cui sono presenti lavoratori atipici l'incidenza della povertà è stimata al 47 Queste considerazioni aiutano a capire l'importanza e l'urgenza che avrebbe avuto un intervento a sostegno di questi lavoratori. Un altro ordine di impegni che il Governo ha completamente disatteso doveva riguardare il recupero del valore reale della cassa integrazione guadagni, che attualmente copre in minima parte la perdita di salario.

Nel provvedimento, avete previsto la possibilità per i lavoratori in cassa integrazione di allungare la durata dei trattamenti loro riservati e addirittura rimpinguarli fino al 100 per cento del salario solo frequentando corsi di formazione forniti dalla stessa impresa presso cui operavano. Speriamo che ciò che tecnicamente chiamate formazione *on the job* non diventi sostanzialmente solo *job*. La misura, inoltre, non migliorerà le opportunità di impiego di quei lavoratori che sono occupati nelle tante imprese in crisi, che probabilmente saranno costrette comunque a chiudere. Lo stesso vale per il sussidio di disoccupazione, che attualmente spetta a tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato assicurati presso l'INPS da almeno due anni, che siano stati licenziati o sospesi dal lavoro, e che copre un valore pari al 60 per cento della retribuzione lorda mensile, per i primi sei mesi, al 50 per cento per il settimo e l'ottavo mese, al 40 per cento per i mesi successivi, per un periodo massimo di un anno. Con questo decreto, il Governo avrebbe invece dovuto implementare le politiche degli ammortizzatori sociali, ricalcolando i costi in base alla realtà economica attuale, per offrire una maggiore equità sociale, attraverso una migliore distribuzione del reddito, a favore delle fasce deboli più esposte alle difficoltà economiche. Le misure sul lavoro sono concentrate nell'articolo 1, e sono - a nostro avviso - da considerarsi assolutamente inefficaci per affrontare la crisi in atto. Un altro dei punti davvero critici è quello della regolarizzazione delle badanti che, per quanto *in extremis*, risolve almeno, anche se solo in parte, le assurde conseguenze del nefasto decreto sulla sicurezza appena votato dal Parlamento, che ha criminalizzato centinaia di migliaia di lavoratori onesti e utili all'economia e alle famiglie, che tuttavia non possono esibire un *curriculum* lavorativo del tutto regolare ai sensi della legge Bossi-Fini. Ci chiediamo, però, se un lavoratore dell'edilizia, dei servizi di pulizia, di cucina o delle fabbriche abbia meno dignità o utilità per la nostra economia. Il provvedimento in esame, anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione anticipa una serie di norme controverse. Mi riferisco al decreto legislativo n. e, soprattutto, all'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego. Certo, una risposta dobbiamo darla alle richieste dell'Unione europea, ma poteva essere realizzata attraverso il meccanismo dei contributi figurativi, riconoscendo il doppio lavoro svolto da chi contemporaneamente ha allevato figli o assistito un parente disabile. Una tale riforma, tra l'altro, avrebbe richiesto un potenziamento dei servizi per l'infanzia e per l'assistenza agli anziani, la cui cura sappiamo essere sempre a carico delle donne. dei Valori aveva presentato un emendamento volto ad incrementare il finanziamento del Fondo per il sostegno della maternità e a prevedere una serie di norme per il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro.

istituzioni pubbliche e dagli Osservatori internazionali, quali la Banca d'Italia, l'ISAE, l'ISTAT, il CNEL e il Fondo monetario emerge una fotografia a tinte molto fosche: in un anno di Governo Berlusconi è diminuito il prodotto interno lordo (meno 5,2 per cento), sono calate le entrate fiscali,

si parla del 118,2 per cento per il prossimo anno: sostanzialmente, in pochi mesi, in meno di un anno, il Governo Berlusconi ha fatto sfumare tutti i sacrifici che, con responsabilità e consapevolezza, il Governo Prodi aveva chiesto agli italiani. È vero che siamo in una situazione di crisi: finalmente lo riconoscete con piena cognizione di causa anche voi.

Voglio porre l'attenzione in modo particolare alle famiglie e agli interventi che proponete per esse. Le famiglie sono abbandonate a loro stesse. In particolare quelle più fragili, che hanno al loro interno un anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente, un soggetto portatore di handicap o affetto da patologia grave o invalidante. È come se queste famiglie subissero una sorta di tradimento. Il decreto contiene la possibilità di regolarizzare le assistenti familiari, chiamate comunemente badanti. L'emersione del lavoro nero è una scelta corretta e condivisa, sicuramente anche da noi, anzi, sostenuta in modo vigoroso e convinto Il punto è che voi proponete la regolarizzazione delle assistenti familiari, delle badanti

è come se non esistessero. Vogliamo tenerli nascosti. Ma se anche ci limitassimo al tema delle assistenti familiari, voglio porvi attenzione particolare, perché questo decreto è inadeguato, non risponde al problema vero del Paese. Sappiamo tutti che la famiglia che assume una assistente familiare non può essere considerata un datore di lavoro. Lo sappiamo Lo sappiamo tutti che c'è una differenza oggettiva tra lavoro di cura alla persona e lavoro di cura della casa, quindi fra badante e colf. Il lavoro delle assistenti familiari è sicuramente un tassello essenziale e irrinunciabile del nostro *welfare* familiare. Si può fingere di non conoscere la realtà in cui viviamo, ma oggi sappiamo che in Italia ci sono 700.000 regolari

Guardando però fra le famiglie che vivono nei nostri paesi, si può ipotizzare che di fronte a una badante regolare, ce ne siano almeno due irregolari. Anzi, si dice che tra le persone che svolgono il lavoro di assistente familiare con regolare permesso di soggiorno, quindi persone entrate con un permesso di soggiorno turistico, il 57 per cento svolge il proprio in nero. Accanto al lavoro nero esiste il lavoro grigio: molte di queste persone denunciano meno ore di quelle effettivamente lavorate. Questa è la fotografia della realtà. È un'Italia fai da te, che ha generato in un anno la bellezza di 10 miliardi di euro. Quindi, non è un dato economico irrilevante non è un dato economico irrilevante ma consistente. È un pezzo della nostra economia e purtroppo - dico purtroppo perché avremmo voluto tutti che la risposta individuata all'interno di questo decreto fosse quella adeguata

che si creassero delle aziende così anomale ed irregolari - quelle sì, erano irregolari - al punto da regolarizzare più persone in contemporanea e creare una sorta di lavoro di lavoro del malaffare e non la regolarizzazione di un lavoro onesto, vero e credibile a sostegno delle nostre famiglie? Purtroppo, questo decreto non affronta tali problemi: avremmo voluto che li affrontasse. Accanto al tema delle assistenti familiari, voglio ricordare un altro aspetto, strettamente connesso e sul quale ieri il Governo, in Commissione,

sui fondi per la non autosufficienza. Cosa avete fatto allora? Avete scelto di non rifinanziare il Fondo per la non autosufficienza. Ieri sera il Governo si è impegnato a riconsiderare

degli anziani e delle persone diversamente abili all'interno delle nostre famiglie: serve una rete di servizi vera, concreta, distribuita su tutto il territorio, che risponda a questi bisogni. Speriamo che tale fondo venga opportunamente e adeguatamente rifinanziato. Altro tema è quello delle giovani coppie.

questa famiglia - lo ricordava anche prima la senatrice Carlino - si trova in estrema difficoltà, perché voi non avete fatto nulla per i lavori atipici e quindi per quei giovani che vogliono far famiglia.

Egli ha usato queste parole: "Penso in modo particolare a come vengono trattate tematiche quali il mercato, l'impresa, la finanza, che in un periodo di crisi come l'attuale sono richiamate ad esprimere al meglio se stesse, facendo ricorso anzitutto al rispetto delle esigenze intrinseche alla loro natura farsi forti delle forme di solidarietà, di retta intenzione e trasparenza, per recuperare quel necessario senso di fiducia senza del quale il mercato, la finanza e la stessa imprenditoria non possono avere futuro. le dinamiche sottese al mercato ed all'impresa, la funzione sociale che svolgono, il valore di genuino apporto al progresso che possiedono nel momento in cui pongono al centro la persona".

vera e piena alla persona umana dentro la società. sono convinto che questo decreto, dal punto di vista dell'efficacia e soprattutto della dignità delle politiche ambientali, segni il punto più basso e la degenerazione più grave da quando è cominciata l'attuale legislatura. Per carità, non ci siamo rassegnati, ma abituati sì, all'evidente anomalia di un Governo e di una maggioranza come quelli che attualmente guidano il nostro Paese, totalmente sordi al tema dell'ambiente e della *green economy*, che in Europa, negli Stati Uniti, e adesso anche in Asia, è ai primi posti dell'agenda politica delle *leadership,* di sinistra come di destra. Del resto, mentre Obama, la Merkel, Sarkozy e Zapatero puntano proprio (non solo nei loro discorsi, ma nei loro atti) loro atti) sull'ambiente e sull'innovazione energetica per rendere più moderne e competitive le loro economie e anche per rafforzare le strategie contro la crisi economica, qui in Italia il nostro Presidente del Consiglio non trova di meglio che dichiarare - lo ha fatto pochi mesi fa che occuparsi delle questioni ambientali in tempi di recessione è come per uno che ha la polmonite andarsi a fare la messa in piega dal parrucchiere. Ha affermato questo tranne poi scoprire, quando si è riunito il G8, che tutti gli altri *leader* con cui era seduto allo stesso tavolo questo tema tutt'altro che marginale e allora ha detto - ma questa è una sua specialità - che gliel'ha insegnato lui. Come si dice a Roma, però, il peggio non è mai morto. Ecco quindi l'articolo 4 del decreto-legge n. 78, la cui conversione in legge stiamo per votare, in cui c'è scritto che d'ora in avanti il Governo potrà decidere che questa o quella infrastruttura energetica non deve più sottostare alle procedure ordinarie di autorizzazione potrà invece essere realizzata in deroga a ogni norma o adempimento ordinari da un commissario nominato dall'Esecutivo. Qualunque infrastruttura energetica, così è detto nel decreto: che sia un impianto eolico o un elettrodotto, una centrale a carbone o una centrale nucleare, un'opera che costa qualche milione di euro o una che ne costa alcuni miliardi.

ci sarà scritto che la scelta delle infrastrutture da sottrarre alle leggi ordinarie dovrà vedere il concerto anche del Ministro dell'ambiente. Ma se questa correzione varrà forse a tacitare le proteste del ministro Prestigiacomo servirà a farle sentire con meno fastidio quanto poco il Governo consideri le sue competenze, essa non cambia però l'essenziale: d'ora in avanti tre o quattro Ministri (sono tre nella versione attuale del decreto, probabilmente diventeranno quattro in quella corretta) potranno decidere, a loro esclusiva discrezione, quali progetti meritino la qualifica di strategici; lascio immaginare con quali rischi di dare spazio a un gigantesco mercato delle vacche, dove vince chi è più amico del potente di turno. Tre o quattro Ministri potranno decidere che - faccio un esempio che non è non è proprio irrealistico - per realizzare una centrale nucleare non servono più quelle fastidiose valutazioni tecniche fatte per assicurare che essa non rappresenti una minaccia per la salute, per l'ambiente e per la sicurezza di chi ci lavora e di chi ci vive intorno. Come ha scritto, non il Partito Democratico, ma il Servizio studi del Senato, non è specificato se questi onnipotenti commissari saranno o meno vincolati al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale. Ma se lo saranno, non si capisce allora in che cosa questa norma accelererà i tempi di realizzazione delle opere; se invece non lo saranno, ciò aprirà evidentemente un contenzioso con la Commissione europea. colleghi della maggioranza, davvero voi pensate che i diritti fondamentali dei cittadini (come il diritto alla salute e il diritto a vivere in un ambiente sano) possano essere ignorati dando poteri assoluti a qualche fiduciario del ministro Scajola? Questa norma non è soltanto iperdirigista (alla faccia del vostro strombazzato federalismo) e non è soltanto evidentemente autoritaria, ma è molto peggio: essa è stupida. Visto che da soli non sapete controllarvi e contenervi, spero che lo faccia l'Europa. Certamente, però, da italiano prima che da parlamentare, io mi vergogno di un Governo e di una maggioranza che su una questione così rilevante per la vita di tutti gli italiani danno risposte tanto indecenti. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che affronta una quantità di temi importantissimi, e ancora una volta non ci viene dato un tempo adeguato per una discussione approfondita. Due giorni scarsi di tempo per la discussione nelle Commissioni riunite e altri due giorni scarsi per l'esame in Aula, con il *diktat* *a priori* che non verranno accettate modifiche. Questo procedere costringe i parlamentari ad un dibattito soffocato dai tempi di conversione aggravati dall'ormai invalsa consuetudine di porre la questione di fiducia che, motivata dall'urgenza dell'approvazione, nasconde la volontà di precludere osservazioni critiche e cambiamenti del testo, privando così di fatto il Parlamento delle proprie prerogative di legislatore. Stiamo discutendo il terzo provvedimento contro la crisi, che ancora non riesce a dare delle risposte soddisfacenti, o meglio, le disposizioni in esso contenute non sembrano affatto sufficienti a far riavviare l'economia e a farci riprendere dalla crisi che stiamo attraversando. Il titolo del provvedimento promette molto più di quello che in realtà contiene. Anche le notizie di stampa e gli annunci riportati dai giornali delle scorse settimane hanno enfatizzato il contenuto del provvedimento facendo credere ai cittadini che contenesse veramente misure in grado di far ripartire l'economia; in realtà le norme contenute sono solo pochi timidi tentativi, sono norme poco chiare che non danno certezza di diritto ma anzi aprono spazi ad interpretazioni diverse per cui, per la corretta applicazione delle stesse, dovremo attendere, anche per questo decreto (come già per molti provvedimenti precedenti), circolari esplicative o altre interpretazioni ufficiali. Riporto solo un esempio: lo scudo fiscale e tutte le interpretazioni sulla materia che circolano. Signora Presidente, mi aspettavo misure più chiare, più precise ed interventi più coraggiosi, sia per quanto riguarda il contenimento della spesa corrente pubblica sia per la riduzione della pressione fiscale che affligge i cittadini e che di fatto purtroppo è aumentata. Mi aspettavo interventi più incisivi per far ripartire gli investimenti e disposizioni più ragionate per il contrasto all'evasione fiscale e non, ancora una volta, un aumento degli obblighi burocratici per i cittadini e un sistema di controlli che, specialmente in certe zone del Paese, ci danno la sensazione di vivere in uno Stato di polizia con soli obblighi e divieti. Soffermandomi su qualche misura contenuta nel provvedimento, voglio sottolineare che ci sono interventi positivi, come ad esempio la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari nuovi. Questa è certamente una buona norma, che però, a mio parere, viene introdotta in un momento sbagliato, perché ci saranno pochissime imprese che avranno le disponibilità finanziarie per farlo. Altre disposizioni positive sono le norme in materia di potenziamento degli ammortizzatori sociali e la riduzione del costo dell'energia per le imprese e le famiglie e le misure per la regolarizzazione delle colf e delle badanti. Accanto a questi, ci sono poi interventi discutibili, come quello diretto ad elevare l'età pensionabile delle donne nel settore pubblico senza affrontare, in modo più approfondito, la politica della famiglia. Infatti, la misura non tiene minimamente conto della diversità che esiste tra l'Italia e gli altri Paesi europei nell'offerta dei servizi sociali a favore delle donne lavoratrici. È questo un tema che ho affrontato molte volte e non solo in quest'Aula. Non è un mistero la carenza di servizi né che gli interventi previsti a favore della maternità e la famiglia siano insufficienti e in forte ritardo. Quindi, la richiesta dell'Unione europea di uniformare l'età pensionabile delle donne a quella degli uomini meritava e merita un approfondimento delle considerazioni sulle donne che lavorano, sulla maternità e sulla famiglia il provvedimento avrebbe dovuto essere accompagnato da interventi di riconoscimento ai fini pensionistici di periodi figurativi di educazione dei figli e assistenza a familiari anziani. Mi auguro che il Governo, attraverso i Ministri responsabili, si faccia presto promotore dei necessari correttivi, integrando la legislazione attuale con disposizioni che migliorino i servizi sociali e che tengano conto del ruolo della donna lavoratrice nella famiglia e del ruolo della donna come madre. Altri interventi, molto discutibili, sono contenuti nell'articolo 9*-bis*, dove, per reperire risorse per l'amministrazione centrale dello Stato, vengono decurtati con effetto retroattivo fondi spettanti alle Regioni, e vengono gravemente disattese le prerogative costituzionali delle autonomie speciali. Per le Regioni a statuto ordinario non è un segnale giusto nella direzione del federalismo fiscale e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il mancato rispetto delle norme dei relativi statuti rappresenta una palese incostituzionalità. Non voglio dilungarmi oltre a commentare altre disposizioni, perché lo faranno ampiamente altri miei colleghi. Concludo quindi rivolgendo al Governo la mia critica, sia per il metodo seguito nell'approvazione del provvedimento, che ha strozzato totalmente il dibattito parlamentare e ha eliminato ogni ipotesi di confronto serio e costruttivo tra le forze politiche su norme che richiedevano una maggiore attenzione, sia per il merito, che non ci convince per le ragioni esposte.

Signora Presidente, dobbiamo pronunciarci sulla richiesta di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in discussione e, nel dichiarare la totale indisponibilità ad accordarla, ritengo di dover richiamare un presupposto fondamentale in tema di fiducia: quello della responsabilità reciproca che ogni atto di fiducia richiede. L'operazione messa in campo dal Governo con il DPEF, con l'ennesimo decreto anticrisi e con un altro decreto che conterrà le correzioni le correzioni obbligate al testo che discutiamo, a causa della necessità di superare le eccezioni dì costituzionalità, è assolutamente censurabile perché difetta totalmente di quel senso di responsabilità a cui è chiamato chiunque amministri *pro tempore* il Paese, in particolare in un momento di crisi così grave. La responsabilità è condizione che correla col tempo, con la condizione adulta: questo provvedimento è irresponsabile perché non si preoccupa degli effetti futuri della crisi, anzi opera scelte che, nel corso del tempo, produrranno proprio gli effetti peggiori, tradendo un principio fondamentale nell'esercizio della responsabilità, che è quello di farsi carico della condizione di chi verrà dopo di noi. irresponsabile continuare pervicacemente a non affrontare in modo strutturale una crisi che è strutturale e non solo congiunturale, come dicono peraltro i dati prodotti dallo stesso Governo nel DPEF appena approvato, che profilano una stagnazione sostanziale ancora per almeno tre anni. È irresponsabile e contraddittorio non farlo adducendo a motivazione l'impossibilità di operare una manovra strutturale ed espansiva come effetto dell'andamento del debito pubblico, che comunque cresce, bruciando risorse accumulate col faticoso e doloroso risanamento dei conti pubblici operato dal Governo Governo precedente. Analogo ragionamento vale per l'adozione frammentata delle misure di contenimento della crisi occupazionale, che si limitano ad una logica di riduzione del danno da disoccupazione, senza occuparsi della necessità di precostituire contestualmente le condizioni per la ripresa dell'occupazione e per il superamento della inaccettabile crasi tra tutelati e non tutelati, o per l'assenza sostanziale di politiche strutturali di sostegno al reddito delle persone e delle famiglie, in relazione alle quali, come purtroppo confermano i dati ISTAT pubblicati ieri, si sta approfondendo il solco tra poveri e poverissimi e ricchi o ricchissimi, tra Sud e Nord, tra donne e uomini, tra giovani e adulti, un solco che il Paese non potrà reggere a lungo.

i supporti forniti da questo strumento sono stati distribuiti a poco più di un terzo dei soggetti potenzialmente stimati fra i destinatari dal Governo al momento del varo; sappiamo, inoltre, che la *social card* è stata fruita prevalentemente dalla popolazione anziana, mentre sempre i dati ISTAT mettono chiaramente in evidenza come le fasce di popolazione maggiormente esposte alla povertà siano le famiglie con un solo reddito e con più figli minori. Quale responsabilità sta esercitando il Governo verso questi bambini, verso questi giovani? Ancora: il Governo affronta la questione dell'età pensionabile delle donne dimostrando assoluta irresponsabilità nei confronti del genere femminile. L'approccio burocratico e il rifiuto al confronto producono una soluzione al problema posto dall'Unione europea che, contraddicendo lo spirito e la lettera della sentenza della Corte di giustizia, amplia, anziché ridurre, la discriminazione di genere e la disparità salariale e confonde (o mistifica) il principio che è sottoposto a quella risoluzione, facendo pagare alle donne i prezzi più pesanti. Ancora una volta, il *welfare* di questo Paese si fa con le risorse delle donne e a danno delle stesse. Non c'è nessun alibi

che l'Italia è in fondo alla lista dei Paesi civili nella propria responsabilità verso lo sviluppo, verso le donne e verso i bambini. Vorrei rapidamente richiamare un altro tema che non posso sottacere. In quest'Aula ieri sera il Ministro ha fatto un'affermazione importante a proposito delle riserve d'oro della Banca d'Italia, dicendo che «l'oro della Banca d'Italia è del popolo italiano». A proposito di responsabilità, si può dire che quelle risorse sono il frutto delle generazioni che hanno prodotto questa ricchezza e delle generazioni che verranno e che ne sono eredi. Proprio per tale ragione, è un patrimonio intergenerazionale e perciò inalienabile e indivisibile: appartiene allo Stato e alla Repubblica e per ciò stesso non è nella disponibilità di nessun Esecutivo, di nessun Governo, nemmeno di questo.

il collega Li Gotti ha già trattato con efficacia, nell'illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità, il nocciolo della contraddizione intrinseca: far votare al Senato la fiducia al Governo su un decreto già sfiduciato dal Governo e far seguire alla votazione l'immediata presentazione di un decreto correttivo. La conversione in legge del decreto anticrisi, già defunto, introduce una sua specifica variante grottesca nel collaudato e ormai abituale schema decreto-legge-maxiemendamento-fiducia, che ormai di fatto ha sequestrato ha sequestrato la potestà legislativa del Parlamento. Ecco in cosa consiste questa variante: si parte dalla legge sulla sicurezza, la nuova legge razziale (come è stata chiamata da illustri commentatori esperti di diritto costituzionale), di diritto costituzionale), in cui si introduce il reato di immigrazione clandestina. Appena approvata la legge si scopre che decine di migliaia di clandestini sono necessari alla società italiana. con l'abituale retorica familistica, ipocrita e tipica del nostro mondo, si riconosce tale necessità solo per le badanti e si fonda così, con una ragione di diseguaglianza anticostituzionale, una differenza tra le badanti e tutti gli altri immigrati impiegati in tutti gli altri lavori socialmente utili. Sono socialmente utili anche quelli, come ha spiegato bene questa mattina il collega Livi Bacci. Sulla base di questa necessità mistificata, cioè salvare qualcuno dentro il mondo degli immigrati clandestini, la legge sicurezza, già pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, resta inapplicata in attesa dell'articolo 1-*ter* del nuovo decreto (quello già sfiduciato), che sospende l'applicazione del nuovo reato solo per le badanti, salvo tornare ad applicarlo in caso di mancata regolarizzazione. si configura irregolare e incostituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Questo sarebbe un saggio, estratto dalla prassi recente del Governo e della maggioranza, di semplificazione normativa, passione di questo Governo al punto tale da dedicarvi un Ministero. C'è da chiedersi che cosa avrà detto il Ministro competente, che credo sia stata ricevuto oggi dal Presidente della Repubblica, in termini di semplificazione normativa. Dei limiti economici di questo provvedimento ha già parlato efficacemente la collega Carlino. Io mi soffermerò su alcuni punti

Evasori fiscali, falsificatori di bilancio, cultori della bancarotta fraudolenta vengono coccolati e incoraggiati a continuare nelle loro specialità disciplinari. riguarda le misure per la lotta ai paradisi fiscali, penso che al G8 molti Capi di Stato avranno manifestato un certo stupore nel veder spingere su questo terreno anche il Presidente del Consiglio italiano, che è notoriamente un esperto di paradisi fiscali. *(Applausi del senatore

Quanto allo scudo fiscale, bisognerebbe ricordare ciò che disse il Fondo monetario internazionale, commentando in un suo rapporto gli effetti dello scudo fiscale applicato in Italia nell'ottobre 2002:

apre un orizzonte di replicazione ininterrotta di condoni e sanatorie. La questione del Ministero dell'ambiente è un buon esempio per giudicare la coerenza del Governo e della maggioranza sia relativamente alla

che creerà. Tale articolo, infatti, reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, qualora ricorrano particolari e non meglio precisate ragioni di urgenza. In questo caso, in nome delle ragioni di urgenza, si stabilisce una tecnica di commissariamento che, su un tema specifico, esclude il Ministero dell'ambiente ed esclude l'esercizio dell'autonomia da parte delle Regioni. Si escludono le Regioni dalla fase di decisione per alcune reti ma non per altre, quasi non esistesse la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia, laddove si prevede - attenzione - che nelle materie di legislazione concorrente spetti alle Regioni la potestà legislativa.

Non solo: su questo terreno, per alcuni punti, viene estromesso e privato di possibilità d'azione lo stesso Ministro dell'ambiente, che infatti non ha mancato di far osservare criticamente la questione. Per quanto

perché la Corte dei conti è un organo indipendente e autonomo che esercita un controllo sulla contabilità dello Stato. Le sue funzioni sono molteplici, ora non le richiamo tutte per non dilungarmi, ma sono ben note all'Aula. Non solo, ma alla Corte dei conti, in materia di risarcimento del danno all'immagine, si richiama la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite civili del 25 giugno 1997, n. 5668, secondo la quale spetta alla Corte dei conti non solo la cognizione del danno erariale, ma anche di quello conseguente alla perdita di prestigio e al grave detrimento dell'immagine della personalità pubblica dello Stato, che seppure non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

italiana - ha rilevato che questa censura, questa sovrapposizione e questa sottomissione della Corte dei conti all'Esecutivo impedirebbero la possibilità delle Corti dei conti regionali di esprimere i propri pareri, perché tutti sarebbero sussunti ad un giudizio delle Sezioni riunite a livello nazionale,

potrebbe immaginare di aprire una questione sul danno all'immagine procurato dal comportamento extraistituzionale del Presidente del Consiglio in relazione a fatti abbastanza sgradevoli, ma che sostanzialmente conviene chiamare per nome e cognome: il giro di donne a pagamento nelle sue residenze. Ora, questo tipo di blocco di possibilità d'azione

La fantasia normativa del Governo e della maggioranza ha trovato dentro questo provvedimento a carico dell'autonomia della Corte dei conti la possibilità di esercitare un intervento protettivo

dire, cioè un momento di depauperamento della possibilità di azione delle Camere elettive. Attraverso questo decreto e gli altri che l'hanno preceduto, sta marciando in Italia una prassi slabbrata, sgangherata e brutta da vedere, che però ha un coerente disegno - orrido - al proprio centro: centro: esautorare in modo sempre più sistematico il libero intendimento delle Camere elettive, per riportare tutta l'azione legislativa nelle mani del Governo, determinando in questa maniera una forma di democrazia che non si sa più nemmeno se sarà tale o una democrazia a sovranità limitata. Dove potrebbe rimanere un minimo di controllo dell'opinione pubblica? Nell'informazione. Ma il nostro è l'unico Paese al mondo in cui il monopolista della comunicazione privata è titolare pieno del potere politico, da dove può controllare anche i mezzi d'informazione pubblici. Allora, per essere consolato qualche volta nella vita, prima di venire qua ho provato a vedere cosa diceva

necessità e inevitabilità di un evento di carattere naturalistico: la cosa deve succedere, non si spiega perché e si racconta così, semplicemente perché fa parte di questa rappresentazione‑finzione,

veramente ai limiti dell'esercizio dei poteri democratici in questo Paese e come non avviene in nessun altro Paese del mondo; devo ribadirlo, perché questa cosa la dovrete sentire fino alla fine di questa legislatura, fino a quando questa storia inverosimile non sarà finita (e sarà sempre troppo tardi quando finirà). È importante ribadire l'azione limitativa delle Camere elettive, il potere sovraordinato del Governo ed il controllo che esso esercita sull'informazione nonché l'abiezione di un'informazione asservita, che non teme di

l'ennesimo decreto-legge sul quale avete posto la fiducia è una nuova prova di forza per nascondere la debolezza dell'Esecutivo ed è l'ulteriore riprova dell'approssimazione e della confusione con la quale si cerca di intervenire nuovamente sull'andamento della crisi economica che sta attanagliando il Paese. Prima di me altri colleghi hanno ripercorso le evidenti contraddizioni e la contestuale inadeguatezza delle misure inserite in questa coperta di Arlecchino che vi ostinate a chiamare misure anticrisi. Si interviene su una miriade di questioni, alcune pertinenti ed altre meno, già affrontate in recentissimi provvedimenti sui quali avete messo la fiducia, ma ancora una volta lo fate in modo scoordinato e senza dare alle norme alcuna finalità strutturale che lasci intravedere una volontà politica di cambiamento in senso riformatore. Si agisce per *spot* ed aggiungendo problemi invece di risolverli, perché questo Governo non è la soluzione bensì, esso stesso, il problema. Mi vorrei soffermare, per rendere più chiaro questo giudizio, su tre questioni che riguardano il sistema infrastrutturale ed i trasporti. La prima riguarda l'incentivazione dell'adeguamento delle strutture aeroportuali. In questa normativa si individuano quali titolari di questo dispositivo i sistemi aeroportuali con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui. È del tutto evidente che si tratta dell'ennesimo capitolo della polarizzazione dello scontro sullo sviluppo del trasporto aereo tra Fiumicino e Milano ed a farne le spese sono altri importanti sistemi aeroportuali (ne cito solo due: Venezia e Catania), che vedono così compromessa la loro capacità di sviluppo e di potenziamento del servizio di trasporto aereo come sistema necessario all'intero Paese e non solo all'asse Roma-Milano. Il riordino del sistema tariffario è un'urgenza per impostare una politica che affronti le principali problematiche connesse a tariffe e servizi. Il lavoro di indagine avviato alla Camera segna però il passo, anche se in questo caso ci si occupa solo di dare risposte a due scali, quelli di Malpensa e Fiumicino, senza la chiara volontà di dare risposte compiute e di riforma del sistema aeroportuale fondamentali per la mobilità interna ed internazionale. La seconda questione riguarda il condono dei debiti iscritti a ruolo, cioè quelli per i quali è stata emessa un'ingiunzione di pagamento derivante da multe elevate entro il 31 dicembre del 2004. È ormai una vostra prerogativa quella di favorire coloro i quali violano la legge e ne escono con agevolazioni e privilegi. Da una parte mostrate la faccia feroce, con provvedimenti all'insegna della galera per tutti, e dall'altra condonate tutti coloro i quali violano la legge e danneggiano la collettività, perché avete il problema di fare cassa e di trovare qualche risorsa per far fronte alla miriade di promesse che continuate a fare agli italiani e che non siete in grado di mantenere. Infine, ricordo il cosiddetto articolo intendete sopprimere gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti. L'aspetto più singolare è che, mentre indicate questa norma come un processo utile a conseguire obiettivi di risparmio di sistema, non ci spiegate in nessuna sede, nonostante ciò sia stato oggetto di ripetute interrogazioni al Senato, alla Camera e in Commissione bicamerale, perché non avete ancora provveduto ad attuare la riforma dei grandi enti previdenziali, dai quali sono previsti risparmi per 3 miliardi di euro. All'attuazione di questa norma è collegata la clausola di un innalzamento delle aliquote contributive. Se tale obiettivo non dovesse essere raggiunto, questa è una delle vere priorità perché non è minimamente ipotizzabile un aumento del costo del lavoro in questa fase di pesante recessione economica, cui la competitività delle nostre imprese deve essere uno degli obiettivi prioritari anche ai fini del mantenimento dell'occupazione. Questa decisione, già presa dal Parlamento e contenuta nella legge finanziaria 2007 (voluta dal Governo Prodi e condivisa dalle parti sociali), è una vera misura anticrisi. aumenta l'efficienza del sistema previdenziale, ne riduce i costi e modernizza una parte non marginale dei servizi della pubblica amministrazione. Voi, invece, preferite, come fa ripetutamente il ministro Brunetta, individuare il pubblico come spreco e non misurarvi con i profondi processi di riforma di cui ci sarebbe bisogno per dare all'Italia gli strumenti, non solo per affrontare la crisi, ma per uscirne con un Paese più forte e più giusto e all'altezza delle sfide che i tempi ci impongono. Con questo provvedimento, si perde ancora una volta la possibilità di definire una strategia agendo sui principali fattori di sviluppo del Paese. Si faccia oggetto di una profonda riforma, consegnando al Parlamento il ruolo che gli è proprio, per un quadro normativo adeguato alle trasformazioni che attraversano l'insieme del nostro sistema economico ed infrastrutturale. puntare sul comparto delle infrastrutture e dei trasporti, appunto, sulle aziende e sugli enti che lo compongono, sul lavoro e sulle competenze che lo devono rendere una leva fondamentale per politiche in grado di invertire il processo di crisi. Purtroppo, invece, soprattutto in questi settori con interventi piegati su piccoli e grandi ricatti territoriali e settoriali. Questo porta a deprimere ancor di più un Paese che meriterebbe un Governo in grado di generali e non alle proprie beghe interne. Il presidente Berlusconi si vanta di non avere mai guidato una maggioranza più forte e coesa di quella che sostiene l'attuale Governo. Se fosse davvero così, avreste il coraggio di affrontare e non di affossare il Parlamento. È per questo che non meritate la fiducia di quella parte del Paese che in noi spera e che ancora ci sostiene.

Durante la discussione generale di questo provvedimento, abbiamo ascoltato la sinistra e l'Italia dei Valori scagliarsi contro il sistema delle banche, quello stesso sistema che, in realtà, loro hanno sempre e sistematicamente sostenuto negli anni in cui sono stati al Governo. Però, dopo aver detto queste cose, vi siete guardati bene dall'appoggiare le disposizioni contenute in questo decreto, fatte inserire grazie alla Lega Nord, che riducono le commissioni delle banche a vantaggio delle imprese e dei cittadini. Noi diciamo che il Governo ha il consenso della gente se governa bene; in questo momento noi abbiamo il consenso della gente perché governiamo bene A dire il vero, questo non è il primo intervento di questa maggioranza contro la crisi, a testimonianza del forte impegno del Governo, che già lo scorso anno ha anticipato gli effetti della recessione mondiale. Infatti, non dimentichiamoci che questa crisi ha origini e responsabilità che varcano i confini nazionali. La verità è che la gente si rende perfettamente conto delle cose. Se ne rende conto perfettamente al Nord, ma se ne rende conto perfettamente anche al Sud: sa che il federalismo è l'unica via d'uscita per poter avere una classe dirigente responsabile, che misura i servizi in funzione della loro qualità e dunque dell'interesse dei cittadini. Abbiamo visto che il Partito del Sud è già stato fatto: le iscrizioni del PD sono percentualmente tutte al Sud, si dovrebbe quindi tornare al nome PDS, però come Partito del Sud! Prima di tutto, si mette finalmente al centro delle politiche industriali ed economiche il sistema delle piccole e medie imprese: non il sistema delle grandi imprese. Si è capito che il sistema delle piccole e medie imprese è l'asse portante della nostra economia, e questa è veramente una cosa positiva. Ancora, si affronta il nodo dei rapporti fra i cittadini, le imprese e le banche. penso alla previsione di un tetto massimo sugli interessi pagati da chi prende i soldi a debito: da domani, dunque, le banche non potranno più fare quello che vogliono. Inoltre, si inserisce una norma che prevede per le banche una moratoria per i pagamenti delle imprese in difficoltà. È un decreto-legge pensato per aiutare la ripresa economica delle imprese, da una parte, e delle famiglie dall'altra. Per primo, c'è il sostegno del lavoro. È un sostegno eccezionale alle famiglie. Si tratta di una misura straordinaria, che dimostra che il Governo non vuole che le aziende licenzino. La Lega Nord non vuole che si lasci a casa nessuno. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Inoltre, si è parlato tanto di scudo fiscale. il fatto che questo tipo di misura è stata introdotta in quasi tutti gli altri Paesi europei, noi ci poniamo una semplice domanda: è meglio far uscire i capitali, come è stato fatto in passato, o farli rientrare? Io penso che oggi sia meglio farli rientrare, perché quei capitali possono e devono servire per fare nuovi capannoni, per acquistare nuovi macchinari, per produrre lavoro; e il lavoro si produce con questo tipo di misure, non con le chiacchiere che voi fate. Hanno già introdotto misure simili la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e l'Ungheria. La Lega Nord vuole però anche maggiore trasparenza e maggior credito da parte del mondo finanziario e delle banche. È prevista inoltre, anche per questo, una rigorosa lotta all'evasione fiscale e ai paradisi fiscali: gli ispettori del fisco avranno i poteri per scovare gli evasori, con la creazione di una vera e propria banca dati antievasione e di scambio di informazioni. Ancora, è stata inserita, grazie all'azione della Lega, una norma che introduce una detassazione per chi Prima di tutto, questa norma è stata costruita in modo tale che serve a finanziare l'acquisto di macchinari e attrezzature prodotti qui da noi. In più, vi è scritto che chi ottiene gli incentivi non può più vendere questi macchinari al di fuori dell'Unione Europea, ovvero non può prendere soldi qui per poi installare gli stabilimenti in Cina. Con un nostro emendamento, è stata introdotta una norma antielusiva: l'agevolazione verrà revocata se i beni oggetto della tassazione saranno venduti all'estero. È un'agevolazione che stimolerà gli investimenti delle piccole e medie imprese, con un naturale aumento dell'occupazione, della produttività e del reddito. Si è voluto poi mettere in regola coloro che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, che potranno essere regolarizzati secondo giuste e precise regole, come sempre abbiamo detto. Lo scopo è quello di tutelare le famiglie che si trovano in condizioni per le quali è necessaria l'assistenza, verificando però caso per caso, in maniera selettiva, le reali necessità. Non è assolutamente una sanatoria, è un volere rispettare le esigenze dei cittadini. Su questo, è stato veramente divertente, questa mattina, sentire parlare la collega Bonino sulle badanti e sulle regolarizzazioni che dovrebbe fare il nostro capogruppo Bricolo: credo invece che dovete badare voi all'ottimo lavoro che lui fa e, con lui, tutta la Lega! Vorrei ricordare un'altra misura molto concreta. Parliamo del sistema delle piccole e medie imprese, degli artigiani, dei commercianti. Vorrei sottolineare che questa norma è stata pensata per una situazione che vivono sulla loro pelle migliaia e migliaia di ambulanti, che nei mercati si vedono sistematicamente scavalcati da quelli che arrivano da fuori, che aprono e chiudono, che non pagano le tasse, che vendono prodotti di bassa qualità, a basso costo, che - come sappiamo - arrivano dalla Cina e dintorni. Ebbene, da oggi in poi, per avere il rinnovo della licenza sarà necessario produrre un certificato di regolarità contributiva. Chi non paga le tasse non avrà più diritto di mettere il banchetto nei mercati e di fare concorrenza sleale a chi dei nostri magari lavora da una vita, pagando sistematicamente le tasse. Inoltre, abbiamo ancora una volta affrontato il tema del Patto di stabilità, che diventa una camicia di forza per gli enti locali. Noi abbiamo previsto che vi sia una possibilità in più per gli enti locali, un ampliamento delle spese che potranno fare i Comuni virtuosi. Anche qui si tratta di fatti e non di parole. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Vi dico che tanti amministratori locali, anche quelli che voi ancora avete, ci chiedono questo e vedono in noi, ancora una volta, l'unico vero e serio interlocutore. Ci saremmo aspettati una atteggiamento diverso, più costruttivo, perché queste norme servono; mentre abbiamo visto una sinistra distante, che non vuole sostenere i bisogni dei nostri lavoratori.

concrete. È un provvedimento che dà una spinta all'economia e mette le imprese nelle condizioni migliori per agganciare la ripresa. Si tratta di interventi positivi, nella direzione voluta dall'apparato produttivo. E su questi fatti, come dicevo prima, ci saremmo aspettati una partecipazione e un appoggio da coloro che sono all'opposizione, perché qui non si tratta di ideologia, si tratta di fatti concreti e di risposte concrete.

Signor Presidente, ieri sera eravamo in quest'Aula, con le Commissioni bilancio e finanze, a discutere fino ad oltre la mezzanotte del decreto anticrisi del Governo. Le senatrici ed i senatori del PD, come sempre e come giusto, hanno fatto il proprio dovere, proprio perché ci divide dal Governo il giudizio sulla crisi; proprio perché non dimentichiamo che tante famiglie al Nord e ancora di più al Sud non potranno partire per le vacanze perché non ne hanno i mezzi; proprio perché sappiamo che molte aziende, piccole e medie, non riapriranno dopo le ferie e molti lavoratori perderanno il posto di lavoro e il reddito; infine, perché siamo donne e uomini di un partito popolare, e le sofferenze e i problemi della nostra gente sono i nostri. Per tutti questi motivi, anche se già ieri aleggiava la richiesta di fiducia, siamo rimasti qui a svolgere il lavoro parlamentare, che poi significa approfondire, tentare di dialogare, tentare di emendare un decreto anticrisi che giudichiamo negativamente, anche se contiene alcune iniziative positive e condivisibili. Non abbiamo fatto niente di più del nostro dovere, ma per la verità l'intera Commissione, opposizione e maggioranza, con il suo lavoro ha dimostrato che tematiche di così grande importanza per le imprese, per le famiglie, per i lavoratori e le lavoratrici, come quelle affrontate dal decreto potevano e dovevano essere trattate attraverso i procedimenti ordinari dell'azione del Parlamento, senza intervenire per la ventitreesima volta con la richiesta di fiducia. A differenza della precedente legislatura, quando la maggioranza aveva numeri risicati, in particolare qui al Senato, questa maggioranza ha un consistente vantaggio numerico. Mi chiedo dunque quale sia la ragione per cui l'imposizione al Parlamento del voto di fiducia è diventata la norma. Che senso ha trattare problemi di questa portata sociale negando al Parlamento le sue prerogative? I problemi che ci pone la crisi pretendono il confronto, che è negato; richiedono la condivisione più larga e il concorso delle opposizioni. Crisi economica, sviluppo, occupazione, povertà, divari Nord-Sud sono i problemi e il futuro dell'Italia e non possono, non debbono, non saranno (non sarebbe possibile), aggrediti positivamente, così come vuole il Governo, mettendo il bavaglio al Parlamento e rendendo irrilevanti le opposizioni. Ogni giorno molti italiani imparano in proprio che non è vero, purtroppo, che la crisi è alle nostre spalle. Questa mattina è stato il Fondo monetario internazionale ad avvertire l'Europa che la ripresa è quantomai incerta e che è del tutto fuori luogo l'ottimismo estivo che vorrebbe vedere soltanto il positivo, e cioè i deboli segnali di rallentamento della recessione. E, guarda caso, il problema più grave che ha indicato il Fondo monetario è proprio quello che diciamo noi da tempo, e cioè che peserà sulla ripresa l'aumento

allarmanti motivi di riflessione che dovrebbero convincere tutti noi a cambiare marcia. Mi riferisco alle statistiche ISTAT sulla povertà, che ci dicono che c'è un aumento spaventoso della povertà, sia quella relativa, così come anche quella assoluta, che cresce del 10 per cento. La povertà è l'indicatore più grave, per un Paese come il nostro, dell'aumento delle diseguaglianze, che sono anche i divari territoriali Nord-Sud, perché parliamo di diseguaglianze concrete tra le persone. L'incidenza della povertà relativa al Sud è superiore di cinque volte alla media del Nord, e sale al 38,8 per cento per le famiglie con figli minori, evidenziando una situazione che in realtà conosciamo da tempo senza però averla mai tenuta nella dovuta considerazione, e cioè quella della forte consistenza in Italia di un'area di minori in pesanti condizioni di disagio. Ecco allora l'importanza che avrebbe avuto tenere al Parlamento, alla sua sovranità e mantenere lì il tema delle misure anticrisi. Non è stato così, ma certo la storia non finisce qui, nemmeno per alcune delle misure anticrisi anticrisi di straordinario rilievo e impatto sociale che sono contenute in questo decreto. Vorrei brevemente riferirmi a tre temi trattati dal è trattato il tema del potenziamento degli ammortizzatori sociali. Non è la prima volta che il Governo interviene e non sarà l'ultima. Ogni volta si introduce un'opportunità in più: in questo caso, la possibilità di utilizzare progetti di formazione e di disporre di trattamenti di sostegno più vicini alla retribuzione ordinaria. Inoltre, la Camera ha introdotto un'ulteriore protezione in materia di ammortizzatori per quei settori che non erano precedentemente coperti dalla cassa integrazione. Il fatto è che il nostro sistema degli ammortizzatori sociali è pieno di buchi. Certamente questo è un problema che non vede insolvente soltanto questo Governo; anche i nostri Governi di centrosinistra avrebbero voluto fare la riforma degli ammortizzatori sociali ma non sono riusciti a farla, a trovare cioè le risorse necessarie per una riforma di carattere universalistico. Ma oggi il tema non è più rinviabile. Questo è quello che diciamo da oltre un anno facendo proposte concrete, appropriate, delle quali siamo convinti e che hanno dato molte prove di validità di fronte agli atti ed ai problemi, e che il Governo non ha mai voluto nemmeno prendere in considerazione e discutere. Così come oggi arriva il momento di guardare a misure necessariamente universalistiche, di contrasto alla povertà, proprio perché l'Italia non può certamente presentarsi in Europa, al di là della retorica, con le misure che finora sono state proposte e predisposte dal Governo - mi riferisco fondamentalmente alla *social card* - cioè misure che si limitano a stigmatizzare la povertà ed i soggetti che fanno ricorso alla carta, dequalificando il nostro sistema di Stato sociale, svuotandolo di ogni ambizione universalistica, che è invece un fondamento per l'affermazione delle tutele, l'esigibilità dei diritti e il superamento di questa crisi. Un secondo tema che voglio sottolineare, su cui sono già intervenuti altri colleghi, a cominciare, stamattina, con efficacia, dall'intervento della senatrice Bonino, è quello della regolarizzazione delle badanti. Una misura che va bene, ma che non basta e che da sola non regge. Prima di tutto resta il *vulnus* inflitto alla civiltà giuridica democratica di un Paese come l'Italia dal decreto sicurezza. Un *vulnus* del quale il nostro Parlamento e tutti noi purtroppo, ahimè, dovremo vergognarci per un certo numero di anni di fronte a tutto il mondo civile perché abbiamo messo fuorilegge tantissimi onesti e preziosi lavoratori immigrati, i quali peraltro contribuiscono alla produzione del PIL con un 10 per cento e ricevono in cambio veramente pochissimo, il 2,7 in termini di assistenza sociale. Oggi, dopo aver scelto di fare la faccia cattiva, si deve correre ai ripari e lo si fa cominciando dalle badanti. In realtà dovremo continuare a farlo per tanti altri lavoratori immigrati e per mille ragioni, non ultimo il fatto che ce lo chiederanno tutte le istituzioni internazionali preposte alla difesa dei diritti. A loro non si potrà rispondere con la faccia cattiva e con il principio dell'egoismo, perché la Repubblica italiana non è la Repubblica padana e neanche la repubblica delle banane. un dovere, innanzitutto quello di aderire ai princìpi costituzionali che sono conformi ai princìpi ed ai diritti umani sanciti da tante Corti internazionali. Per ultimo, e concludo, due battute sull'aumento dell'età pensionabile per le donne nella pubblica amministrazione. La sentenza della Corte di giustizia richiede parità, ma non chiede mica la lesione dei diritti acquisiti per una specifica generazione di donne. Mi riferisco proprio a quelle che dovrebbero andare in pensione a partire dal 2015 perché hanno maturato il requisito, alle quali si riserva il danno e la beffa. beffa. Non capisco la ragione per la quale proprio dal risparmio previdenziale realizzato su quel gruppo di lavoratrici dovrebbe venire il contributo al fondo per la non autosufficienza, quando invece è ben chiaro che la disabilità è una condizione fortemente tutelata dall'articolo 3 della nostra Costituzione, laddove si dice che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale... ». Quindi, in quanto tale,

con la dubbia solidarietà a danni di un gruppo di lavoratrici. Alla Corte si deve rispondere con misure coerenti e non improvvisate. Per questo serve un altro modo ed una larga condivisione, in particolare per quanto riguarda il patto sociale, perché parliamo di lavoratori che contribuiscono alla pensione con i loro contributi, non soltanto pubblici. Serve un dialogo ed una concertazione con le parti sociali. Infine, la parità si può fare, a nostro avviso, e si dovrebbe fare non necessariamente penalizzando le donne, ma garantendo libertà di scelta e flessibilità per uomini e donne, senza inutili forzature, peraltro in aperta contraddizione con altre misure contenute in questo decreto, come quella che prevede la pensionabilità nella pubblica amministrazione con 40 anni di contribuzione figurativa, sulla base della cessazione unilaterale del rapporto di lavoro. Pertanto, si potrebbe verificare il caso veramente grottesco, per cui, da una parte, si chiede ad una donna di restare a lavorare nella pubblica amministrazione fino a 65 anni e contemporaneamente la si caccia, magari perché non gradita, sulla base appunto delle norme introdotte in questo decreto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sin dal suo insediamento il presidente Berlusconi e il Governo si sono adoperati per sostenere il sistema economico e finanziario del nostro Paese. Una volontà, questa, che è stata indotta e fortemente condizionata dalla crisi economica mondiale, la cui genesi e le cui responsabilità varcano i nostri confini, e che ha provocato il poderoso rallentamento dell'economia e l'inversione generalizzata del PIL in tutti i Paesi industrializzati. Una crisi rispetto alla quale i più importanti Governi del mondo si sono dovuti loro malgrado confrontare, mettendo a frutto strategie volte, da un lato, al contenimento degli effetti e, dall'altro, ad una possibile inversione di tendenza. In questi mesi l'azione del presidente Berlusconi è stata quella di cercare di garantire condizioni di stabilità per la finanza pubblica, salvaguardando il sistema creditizio, il risparmio delle famiglie, sostenendo i redditi ed i consumi. Il Governo, nonostante la presenza di forti vincoli di bilancio, ha fronteggiato la recessione con una condotta duale, operando sia con misure di stimolo fiscale sia con misure di supporto finanziario. Purtroppo, ahimè, i tempi duri - lo sappiamo tutti - non sono ancora finiti. E se oggi gli Stati Uniti vedono un presidente Obama particolarmente ottimista (che esalta i suoi sforzi, le misure anticrisi approvate per risollevare l'economia e forse intravede la fine della crisi) e se oggi anche in Italia giungono alcuni segnali che indicano una decelerazione della crisi (torna a crescere il numero delle imprese, la produzione industriale sta consolidando le sue posizioni), colleghi, forse siamo solo al giro di boa. I dati sulla disoccupazione e sulla povertà non possono di fatto farci E per questo, proprio in relazione al protrarsi della gravità della situazione economica-finanziaria interna ed internazionale trova giustificazione l'adozione, a ridosso della pausa estiva, di questo provvedimento d'urgenza, pur necessitando delle modifiche e dei correttivi che saranno varati nell'immediato dal Consiglio dei ministri. Colleghi, il decreto-legge n. 78 del 2009 è senza ombra di dubbio un provvedimento importante, che giunge alla fine di un periodo durante il quale la struttura produttiva del Paese è stata sotto le bordate della crisi economica. Un provvedimento che si pone in continuità con gli altri interventi economici messi in campo dal Governo Berlusconi, nell'ottica di una azione a piccoli passi, una politica di interventi puntuali e precisi, che di volta in volta cercano di mitigare e risollevare la non certo appassionante situazione del Paese. Questo, infatti non è ovviamente il primo intervento anticrisi di questa maggioranza, proprio a testimoniare, a certificare l'impegno dell'Esecutivo in questa direzione. Non una politica di spizzichi e bocconi, senatrice Leddi, ma una serie di interventi, una successione ininterrotta di azioni mirate, che con specificità sono intervenute per ridare slancio all'economia, alle imprese, ai cittadini, alle famiglie. Penso all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, alla rinegoziazione dei mutui, ai *bonus* alle famiglie, alla detassazione degli straordinari, all'IVA per cassa, alla revisione degli studi di settore. L'Esecutivo, in poco più di un anno di governo, è intervenuto tempestivamente, ora in difesa delle famiglie in difficoltà, ora delle imprese, ora sostenendo i comparti produttivi strategici, ora assicurando il trattamento di integrazione salariale anche per quei lavoratori che fino ad oggi ne erano sprovvisti, ma sempre garantendo per ogni azione un equilibrio tra entrate e uscite: interventi portati avanti senza dover mai aumentare le tasse e ridurre la spesa sociale. Ora è inevitabile intervenire di nuovo ed è inevitabile farlo oggi. Certo, colleghi, per risolvere le emergenze e affrontare l'evolversi della crisi economica si è fatto spesso ricorso allo strumento del decreto-legge si è spesso posta la questione di fiducia, come in questo caso, ma senza commettere mai l'errore di mortificare e sminuire le prerogative del Parlamento. A fronte della grave situazione in atto c'è la necessità di legiferare in tempi rapidi e dare risposte immediate alle esigenze dei cittadini. Il decreto-legge oggi in discussione, che ha le caratteristiche di coerenza e di uniformità rispetto alle scelte adottate sino ad oggi dall'Esecutivo, si pone l'ambizioso ma reale obiettivo di aiutare, da un lato la ripresa dell'economia e delle nostre imprese e dall'altro le famiglie italiane. Il testo contiene infatti significative prescrizioni in materia di fiscalità agevolata per gli investimenti delle imprese, di allentamento del Patto di stabilità per gli enti locali, di ammortizzatori sociali e di incentivi all'occupazione. altresì misure per la regolarizzazione di colf e badanti e di coloro - sono migliaia in Italia - che svolgono attività di assistenza e sostegno alle famiglie, agli anziani e a tutte quelle persone che si trovano nelle condizioni di non autosufficienza. Il decreto-legge contempla poi importanti disposizioni di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, all'emergenza abitativa, di rafforzamento dei meccanismi di tutela dei clienti dei servizi bancari di contrasto ai paradisi fiscali. Esso stabilisce anche norme di semplificazione per gli interventi di produzione e distribuzione di energia; allunga la durata della cassa integrazione straordinaria e, allo stesso tempo, consente al lavoratore percettore di cassa integrazione guadagni di ricevere in un'unica soluzione (anziché mese per mese) l'ammontare spettantegli, così da avere un capitale iniziale per poter magari avviare una propria attività. questo solo per citare alcuni degli interventi contemplati nel disposto normativo che stiamo valutando. Si tratta di una sommatoria di interventi che, se considerati singolarmente, potrebbero ad una frettolosa analisi apparire di poco conto, in realtà tutta la loro efficacia e portata se si considera il provvedimento nel suo insieme e congiuntamente alla strategia organica messa in campo in questi mesi dal Governo. Certo, il lavoro che ci aspetta, e che aspetta il Governo, per ridare fiducia e slancio all'Italia non è certamente esaurito: occorrono impegno e responsabilità da parte di tutti noi per consentire al Paese di uscire da quella spirale negativa in cui è precipitata la nostra economia. Concludendo, signor Presidente, è evidente al di là di ogni ragionevole dubbio che la portata del testo è significativa e quanto mai rilevante, soprattutto alla luce della difficile congiuntura che investe il Paese, della condizione di ristrettezza delle risorse, del debito pubblico e degli eventi contingenti che hanno fatto da cornice alla stesura del provvedimento. Colleghi, abbiamo la responsabilità di dare risposte al nostro sistema economico, e questo è un provvedimento che contempla numerosi interventi destinati a dare una spinta all'apparato produttivo italiano e a mettere le nostre imprese nelle condizioni di agganciare la ripresa. Certo - lo ripeto - si poteva fare senz'altro di più. Ho ascoltato con attenzione molte delle rivendicazioni giunte dai banchi dell'opposizione, alcune frutto anche di plausibili ragionamenti politici, allo stato attuale, non è accettabile per il Paese continuare a portare avanti un'azione contro, comunque, o battersi per vedere accolto un ragionamento esclusivamente localistico. Dobbiamo pensare al sistema nella sua interezza, come ad una macchina in cui tutti gli ingranaggi - le nostre Regioni e le singole realtà - concorrano congiuntamente a far muovere e crescere il Paese. Ognuno di noi in quest'Aula potrebbe certamente rivendicare qualcosa; io potrei farlo per la mia Regione,

così come è necessario un piano per il rilancio del Sud e le opere strategiche per il Mezzogiorno: interventi che il Governo realizzerà perché inseriti all'interno di una logica generale che investe tutto il sistema Paese, nella quale mi riconosco.

certamente nel dibattito su un decreto anticrisi non mi aspettavo di udire parole ottimistiche, né temi e toni improntati al trionfalismo, ma al trionfalismo, ma francamente nemmeno di assistere ad una serie di interventi così pesanti, con orizzonti bui, disastri globali ed impossibilità di risorgere. Forse un po' di esagerazione c'è; dopotutto, questo è il ruolo che qui ciascuno di noi esercita. Dovessi accettare questo tipo di scenario, non avrei nemmeno il coraggio di cominciare a parlare per innestare su una crisi congiunturale un problema di difficoltà endemica e cronica

In fondo, poi, è davvero molto tempo che non parliamo di queste problematiche, non soltanto di montagna ma in genere di territori svantaggiati. Non lo faccio certo con lo spirito di chi aggiunge, come dicevo, miseria a miseria, ma come promemoria e come richiamo al Governo affinché non si dimentichi che, al di là di là delle congiunture, vi sono problemi che sono da considerare soltanto in *standby*, in attesa cioè di essere ripresi. Le politiche per la montagna da sempre sono la Cenerentola delle politiche territoriali, regionali e nazionali, anche se la montagna in Italia rappresenta oltre il 50 per cento delle amministrazioni comunali; ma purtroppo in montagna vive soltanto il 12 per cento della cittadinanza italiana, quindi è una massa critica non molto interessante nemmeno sotto il profilo politico-elettoralistico, anche se la montagna da sola produce circa il 20 per cento del PIL, ottenuto, per giunta, in condizioni di reale difficoltà.

come questo, ha sempre dimostrato di avere una reattività maggiore rispetto ai centri urbani, una capacità di organizzarsi,

tutti i valori risultano amplificati, nel bene e nel male; quindi anche una crisi come l'attuale nelle zone montane si è manifestata in maniera particolarmente pesante, soprattutto perché viene ad innestarsi su un sistema sociale ed economico già di per sé fragile e provato da molte altre crisi e difficoltà endemiche. In questo momento le due grandi risorse della montagna, l'agricoltura e il turismo, sono a dir poco in ginocchio (non dico prostrate per non offendere coloro che si stanno impegnando).

Per quanto riguarda il turismo, si è appena chiusa la stagione invernale, con un risultato che è stato definito dalle associazioni di categoria di pura sopravvivenza: nessun investimento, nessun intervento particolare, pare che nemmeno gli impianti di risalita possano essere rimessi a posto e tanto meno gli impianti alberghieri.

l'economia e l'equilibrio generale rischiano di crollare per molto tempo. Aumenta, come tutti sappiamo, il turismo detto mordi e fuggi: le famiglie partono al mattino con lo zaino pieno di panini, e tornano alla sera, e per giunta si lasciano come *souvenir* tutti i rifiuti sul territorio; quindi i Comuni devono anche provvedere a ripulire prati, sentieri e strade. Sembra che certi ristoranti, quelli veri e propri, siano ormai riservati a pochi intimi, ma anche le pizzerie, che erano il rifugio tradizionale delle famiglie, a costo di dividere una pizza tra tre bambini, rappresentano

quella gente che decide ancora di rimanere a vivere lassù o che ci va a vivere in cerca di un'occupazione. Questo sviluppo è anche utile per salvare testimonianze storiche e culturali, patrimoni ambientali che le multinazionali del grande turismo, quelle attività dei grandi villaggi turistici, non solo non tutelano, ma spesso anzi deturpano.

della montagna», che lancia un autentico appello per correre ai ripari finché si è in tempo. Questo documento sostiene tra l'altro che è arrivato il momento d'invertire il processo di urbanizzazione, facendo della montagna e dello spazio rurale i fattori di un nuovo sviluppo dell'Italia. La strategia di riequilibrio territoriale dello sviluppo non deve essere confusa con le tradizionali logiche di sostegno ai territori in difficoltà; al contrario, si tratta di guardare alla montagna e allo spazio rurale come straordinarie risorse per il rilancio di processi di crescita nazionale basati sulle filiere più innovative e promettenti anche dal punto di vista economico.

prodotti tipici che nascono da soli e non occorre produrli con sistemi biologici, ma è sufficiente rispettare il sistema della natura. Questo è già presente in montagna, e infatti sono queste le fonti di sopravvivenza di cui parlavo prima.

L'imprenditoria è fondata sempre sul coraggio, ma anche su molta individualità, sull'orgoglio - come dicevo prima - di potercela fare anche da soli. Questo, tuttavia, non basta più e bisogna mettere a frutto qualche misura particolare; proverò quindi a formulare qualche proposta concreta:

una terza proposta potrebbe consistere in una deroga dal regime degli aiuti di Stato e dalle regole della concorrenza per consentire aiuti anche di sistema. Inoltre, sarebbero utili nuove norme per l'assunzione del personale stagionale, incentivi per la multifunzionalità e le professioni tipiche della montagna, come la

un aspetto delicato: è necessario anche guardare con serenità ed obiettività al prezioso ruolo che esercitano alcuni enti intermedi sovracomunali nelle zone più periferiche, a beneficio soprattutto dei Comuni più piccoli. Questi enti sovracomunali provvedono a fare qualcosa che i piccoli Comuni da soli non riuscirebbero a fare, compresi servizi di vitale importanza. La caccia alle streghe che si è innescata non molto tempo fa a proposito della riforma delle comunità montane ha finito per coinvolgere, accanto a realtà che in effetti andavano soppresse o modificate, anche molte altre piccole realtà che sono necessarie e che vanno invece salvaguardate. Bisogna oggi guardare anche con un occhio diverso e più sereno al tema delle spese, che potrebbero essere rivisitate con maggiore realismo e conoscenza anche delle realtà territoriali, senza demagogie persecutorie. Questo è un ruolo che spetta chiaramente al Governo con il contributo delle Regioni. Purtroppo, è qui che l'appello diventa difficile, in quanto il tema montagna e specificità ancora una volta ha tanto il colore dell'abito di Cenerentola. Nella precedente legislatura si è visto purtroppo un record negativo, in termini di disinteresse, da parte dall'allora Ministro per le Regioni con delega per la montagna: non solo in due anni non ha mai assunto una iniziativa a favore della montagna, ma ha demolito quanto era stato fatto dal suo predecessore. L'attuale Ministro per le politiche regionali e la montagna - va detto in maniera esplicita - a sua volta non è riuscito a produrre alcun intervento che vada direttamente nella direzione della montagna, preso dalla contingenza imprevedibile di questa crisi e anche sommerso dagli impegni

credere a coloro che già intravedono in fondo al tunnel uno spiraglio di luce, se questo spiraglio diventerà un faro e poi finalmente luce piena e la crisi sarà superata, spero solo che potremo tornare ad occuparci delle normali difficoltà che

all'esaurimento. Abbiamo sentito parlare di Repubblica della Padania, del resto ingenerosamente abbinata alla repubblica delle banane. questi discorsi anche quando venite nelle nostre terre a chiedere voti in campagna elettorale? Vedreste come vi tratterebbero i nostri conterranei. Abbiamo sentito parlare di piano Sud che non c'entra niente con questo provvedimento, di soldi veri o falsi e di soldi che non ci sarebbero, della paura che il piano Sud possa diventare il piano Berlusconi, prendendo il nome del *Premier*.

com'è complessivamente. Infatti, oggi uno Stato dovrebbe innanzi tutto intervenire massicciamente in tutti i settori economici che sono in difficoltà per dare loro un po' di ossigeno e poi dovrebbe incrementare la spesa pubblica per mettere

aiutare le piccole aziende municipalizzate, che per stare sul mercato dovevano inevitabilmente aumentare i costi, ad avere oneri amministrativi minori, per consentire loro di erogare buoni servizi a costi più bassi. A noi sembra assai interessante quella

enti locali virtuosi che hanno somme accantonate e hanno bisogno di fare investimenti, ma per le norme restrittive dei patti di stabilità non possono farlo. Svincoliamo non chi ha le casse in dissesto, ma chi ha tutti i conti in ordine i soldi da parte e nemmeno si indebita, cosicché possa mettere in moto grosse

perché noi legislatori pensavamo di essere le persone più acute del Paese e abbiamo approvato importanti protocolli e rigidi disciplinari per stabilire ciò che si può portare in discarica, elencando, elemento per elemento e quantità per quantità, ciò che è pericoloso ed eventualmente nocivo.

la tracciabilità del rifiuto, ovunque esso finisca. È stato ingenerosamente criticato il passaggio tendente ad

non ha accettato il deliberato delle Commissioni della Camera. Questo è un fatto di una gravità inaudita. Il mancato rispetto del Parlamento, come diceva il collega Pardi, è la caratteristica della vostra azione politica.

al di là del bicameralismo o meno, si fonda sull'importanza del Parlamento. Questo esproprio deve finire. Si espropria il Parlamento giorno per giorno e ve lo dimostrerò, almeno

issando bandiere, utilizzando la sofferenza per esaltare una politica che non c'è per quanto riguarda il terremoto. L'uguaglianza è nelle norme. Noi ci faremo promotori, signor Presidente

Il presidente della Regione ha un ruolo di programmazione e deve mantenerlo, ma il commissario deve tutelare i LEA, i diritti della gente, non può essere colui che ha portato allo sfascio la sanità, soprattutto nella mia Regione,

Credo che questo Governo debba ridare dignità a questi lavoratori che stanno al Nord e devono avere tutta la dignità possibile per esercitare il proprio ruolo.

in queste ore, in cui milioni di italiani stanno andando in vacanza, per fortuna, siamo impegnati in un dibattito che ha qualcosa di surreale, e non perché stiamo parlando di crisi, ma per come il Governo ha imposto di discuterne a questo Parlamento. Ci rendiamo conto, colleghi, che

di che cosa dobbiamo mai discutere? È molto mortificante, per noi,

non posso incidere su quei disegni di legge che li riguardano direttamente, e non posso farlo perché la politica voluta dal nostro presidente del Consiglio Berlusconi è una politica populista, che vuole ridurre questo Parlamento a poco più di un orpello. Così come considera ininfluenti i sindacati, un fastidio i partiti e probabilmente, in cuor suo, anche inutili le elezioni democratiche in questo Paese. Vedete, colleghi, al contrario del mio amico senatore Morando, sono un convinto fautore del bicameralismo, che va sicuramente modificato velocemente i Regolamenti parlamentari e questo Parlamento deve recuperare efficienza, in questo ramo come nell'altro, ma penso che il bicameralismo preservi fino in fondo la capacità di democrazia della nostra Repubblica e la capacità del Parlamento di rappresentare gli interessi di questo Paese.

Ebbene, in Commissione sanità siamo unanimemente convinti che il medico non possa essere considerato meramente un ingranaggio della nostra burocrazia, il dirigente medico debba essere considerato come il primario e che sia discriminante considerarlo diversamente dal primario, che invece non viene rottamato, insieme ai magistrati e ai professori universitari, inserendo in modo surrettizio l'idea che esistano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B

sul commissariamento, probabilmente giusto in alcune Regioni come la Campania, il Molise e la Calabria. Ma basta una visione burocratica di commissariamento o non ci vuole forse una politica più strutturata, di ampio respiro per la sanità di questo Paese? Forse i tagli trasversali non bastano. Dobbiamo avere l'idea di recuperare efficienza ed efficacia nel nostro sistema sanitario, renderlo più uguale in tutte le parti del Paese. Allora un provvedimento che doveva rendere più giusto, più uguale il Paese si trasforma invece in un atto di autorità,

L'universalismo o c'è o non c'é, non può essere selettivo perché, se è selettivo, voglio capire nei confronti di chi. Siccome stiamo facendo tagli trasversali indiscriminati, probabilmente a rimetterci saranno i soliti cittadini, quelli che oggi pagano i *ticket* e che domani ne pagheranno di più, sempre di più, anche quelli più deboli.

avevo fatto riferimento ad un parere della Giunta per il Regolamento del Senato che, in merito alla fiducia, si esprimeva con la richiesta di fiducia il Governo condiziona espressamente all'approvazione di un testo la propria sopravvivenza. Oggi noi sappiamo che il Governo lega la propria sopravvivenza ad un testo che invece non vuole più, perché lo sta cambiando.

Ovviamente la questione della fiducia, che è cornice della discussione, sposta l'oggetto del nostro esame, che si riduce esclusivamente a scampoli di valutazione su un provvedimento comunque complesso. Tuttavia anche

Sentite bene che cosa stiamo approvando: «L'azione per il recupero del danno da immagine

«Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma» - ossia quelle che ho appena letto «è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento». Ossia, lo scopo dell'accertamento viene posto invece quale presupposto per poter fare l'accertamento a pena di nullità. L'atto istruttorio L'atto istruttorio deve essere assistito dal presupposto di un fatto che invece l'atto istruttorio è destinato ad accertare, perché il requisito del dolo o colpa grave deve assistere e precedere il compimento dell'atto istruttorio a pena di nullità, rilevabile in qualsiasi stato e grado, fatta valere da chiunque, in qualunque momento, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di 30 giorni. Ciò significa che qui allora non si tratta di ancorare all'esistenza del danno per colpa grave o dolo l'azione di responsabilità, perché anche l'accertamento dell'eventuale danno per dolo o colpa grave viene reso reso impossibile dal momento che ciò che si vuole accertare deve essere invece già accertato. Questa è ipocrisia bella e buona. significa non accertare. Significa che le procure distrettuali contabili non potranno accertare se esiste il dolo o la colpa grave, perché devono essere già accertati, essendo questo un presupposto. Questa è una grande forma di ipocrisia per dire che la procura contabile non deve più fare accertamenti. Sullo scudo fiscale, al comma 4 dell'articolo 13‑*bis*, si richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 350 del 2001, che a sua volta rinvia all'applicazione del decreto‑legge n. 143 del 1991, che è norma abrogata, cioè si rinvia ad una procedura normativa che non fa parte del nostro ordinamento. Sul problema della regolarizzazione degli irregolari, ancora ricordiamo l'alto insegnamento giuridico del ministro Maroni,

«Anche uno studente al primo anno di università sa che questa norma non si applica agli irregolari presenti nel nostro Paese». Ci fece una lezione di diritto, ci chiamò tutti ignoranti. Poi qualcuno gli spiegò che il reato di soggiorno irregolare è un reato permanente: non posso essere punito per ieri, quando non c'era la fattispecie di reato, posso essere punito per l'oggi, nel momento in cui viene introdotta la fattispecie di reato. E allora, dopo che abbiamo assistito a queste dotte disquisizioni giuridiche, siamo arrivati - a me dispiace non ci sia il sottosegretario Caliendo, che è un giurista

che i reati di soggiorno e ingresso illegale vengano dichiarati estinti, quando invece la possibilità era quella di dichiarare la non procedibilità per il sopraggiungere di una diversa condizione. Il prevedere invece l'estinzione del reato significa introdurre un'amnistia che, ai sensi dell'articolo 79 della nostra Costituzione, prevede una maggioranza qualificata dei due terzi, oltre la che è stata già denunziata più volte, dell'articolo 3 della Costituzione. La medesima cosa riguarda l'estinzione di fatto dei reati di di esportazione di capitale, mancata denunzia, infedele denunzia e omessa dichiarazione. vengono estinti di fatto e diventa quindi anche questa un'amnistia, non potendo essere utilizzabile nei confronti del contribuente l'accertamento derivante dal rientro dei capitali detenuti all'estero.

nella normativa sulla distribuzione e sulla produzione di energia si prevede la competenza esclusiva dello Stato quando la stessa, ai sensi dal comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è materia concorrente. Vengono escluse le Regioni, sottraendosi alle stesse la competenza legislativa perché, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117, nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa.

scampoli di valutazione che fanno capire come sicuramente i correttivi che verranno introdotti domani dal Governo cambieranno qualche cosa, ma rimangono la profonda ipocrisia di questo provvedimento e la profonda incostituzionalità dello stesso.

il diritto del Parlamento a svolgere le sue competenze legislative e il diritto del Governo a dare risposte all'altezza dei tempi e dell'emergenza. Credo che anche l'opposizione debba convenire sul fatto che avanza una Costituzione materiale, che si è imposta sia in questa legislatura che in quella precedente, che consiglierebbe alle Camere di rivedere i propri Regolamenti parlamentari per assicurare certezza di tempi al Governo e la via di una equilibrata democrazia decidente attesa dal Paese. Tutto qui. Per questo è eccessivo, credo, parlare di rappresentanza violentata oppure di Parlamento imbavagliato (queste le espressioni usate qui e lì). Non escludendo, per onestà, che il ruolo del Parlamento e l'esercizio delle sue prerogative (in questo quadro mutato) esista in tutta la sua significanza costituzionale. Per venire al merito del provvedimento, l'emanazione di otto decreti, con questo, in materia economica è la conferma che il Governo ha provato a replicare e a contrastare, con equilibrio e prudenza, i problemi indotti da una crisi la cui portata si è via via manifestata ed i cui effetti non erano, peraltro, prevedibili. Il Governo, anche con questo ultimo provvedimento, prova a dare risposte alle parti sociali più direttamente colpite, con le misure di allargamento e di potenziamento degli ammortizzatori sociali, implementando un'azione interessante sotto il profilo sociale e sperimentando progetti di formazione-lavoro che puntano a non disperdere lo straordinario capitale di competenze che si è formato a ridosso delle nostre aziende, in attesa di una possibile ripresa delle attività produttive. Un nuovo *welfare* che fa degli ammortizzatori anche una possibile opportunità per esplorare nuove strade di reimpiego per i lavoratori colpiti dalla crisi della propria azienda, oppure per acquisire nuove competenze professionali. Come pure, l'aver assunto il tema della regolarizzazione di colf e badanti risulta un atto di regolarizzazione di persone impegnate nella cura delle nostre famiglie e nello stesso tempo smentisce l'idea, agitata anche questa sera, di un Governo ostile per principio al contributo di tanti stranieri che invece collaborano alla vita delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Ed ancora, gli incentivi fiscali per società e imprese, per la per la loro capitalizzazione e per una ripresa degli investimenti nelle attrezzature non fanno parte di una manovra anticiclica, ma finalizzata a preparare anche la ripresa che si attende, dando più consistenza al patrimonio delle aziende e sostenendo un processo di innovazione. Inoltre, per le imprese non è da sottovalutare l'intesa con il sistema bancario per ottenere una moratoria sui debiti, condizioni di costo meno onerose sui servizi di credito ed anche un più facile e più ampio accesso al credito stesso. Questa consapevolezza dell'esigenza di non far mancare il credito al sistema delle imprese in un momento delicato e di crisi ha portato il Governo ad inserire in questo provvedimento le norme finalizzate alla velocizzazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione per i debiti accumulati negli anni da parte degli enti pubblici. sempre nella prospettiva di premiare la virtuosità degli enti locali, che hanno concorso a preservare il Patto di stabilità del nostro Paese e nello stesso tempo per corrispondere ad una esigenza di ripresa degli investimenti, si deve interpretare la misura di attenuazione del Patto di stabilità per gli enti locali stessi, con l'esclusione dal vincolo di alcuni pagamenti per investimenti in conto capitale. La manovra, che ammonta a 12,5 miliardi di euro, si

*(PdL)*. Noi crediamo che il Governo debba proseguire sulla via del rigore, della qualificazione della spesa, della sua finalizzazione.

sapendo imporre anche un'azione di coordinamento tra i programmi di spesa nelle Regioni del Sud che in questi anni è mancata, a vantaggio spesso di cicli di spesa improduttivi che hanno alimentato più reti di consenso che infrastrutture di sviluppo. Proprio a partire dal Mezzogiorno,

Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi rivolgo agli onorevoli colleghi presenti. Ci ritroviamo ancora una volta in quest'Aula, tra l'altro esautorata dalle prerogative che la Carta costituzionale le attribuisce, a varare un provvedimento anticrisi nel quale l'agricoltura continua a giocare il ruolo di una semplice comparsa. Mi scuseranno i presenti se parlerò solo di questo settore, di cui non vi è traccia in questo provvedimento anticrisi. Stiamo parlando di un comparto che rappresenta il 16 per cento delle imprese italiane vale circa 220 miliardi di euro, ma di cui questo Governo, in un momento in cui l'intera economia del Paese è stremata dai riflessi di un quadro congiunturale pesantemente negativo, non si occupa minimamente, manifestando così, oltre che un perdurante disinteresse, anche una notevole dose di miopia. Infatti, dimenticare le difficoltà ed i rischi che sta affrontando il comparto agricolo e le ricadute che questi hanno sull'industria alimentare, sull'occupazione e sui consumi dei cittadini, dimostra una superficialità e una debolezza strategica preoccupanti. Recenti indagini testimoniano come in molte aree del mondo i nostri prodotti alimentari rappresentino la prima categoria merceologica che richiama alla mente il *made in Italy*; fatto, questo, che testimonia la necessità di approntare una strategia volta al rafforzamento del sistema agroalimentare italiano che abbia una prospettiva di medio-lungo termine, che sappia attivare politiche dedicate alla crescita strutturale, organizzativa, all'integrazione, agli strumenti di difesa dai rischi, tanto più che negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni di volatilità dei prezzi mai sperimentati prima che mettono seriamente a repentaglio la sopravvivenza di grosse porzioni del tessuto imprenditoriale. Nonostante queste premesse, nel corso degli ultimi dodici mesi di legislatura il Governo ha mostrato completamente l'incapacità di approntare una politica di rilancio del settore: rincorre il quotidiano e si occupa dell'esistente, come se la crisi non l'avesse neppure sfiorato. Considerate che in altri Paesi come la Francia si sono stanziati 250 miliardi di euro per il rilancio del comparto agricolo e che Paesi come la Germania e la Spagna hanno avviato riforme importanti per ridare slancio all'agricoltura

Quando deciderete di occuparvi delle preoccupazioni degli imprenditori del settore, molti dei quali vedono a rischio la tenuta delle proprie aziende e il mantenimento dei livelli occupazionali? Quando smetterete di guardare con noncuranza dati sempre più allarmanti che ci parlano di migliaia di imprese agricole destinate a chiudere a causa di costi produttivi e oneri sociali praticamente raddoppiati? Mi chiedo: quando il Presidente del Consiglio deciderà di onorare la sua promessa, fatta alla presenza di 15.000 agricoltori all'Assemblea nazionale di Coldiretti, sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà, di cui ancora non vi è traccia in questo provvedimento? Mi rendo conto che parlare dall'affidabilità della parola di quest'uomo può far sorridere, ma vi assicuro, onorevoli colleghi, che gli agricoltori non sorridono affatto di fronte ai costi di produzione (concimi e benzina in testa) praticamente raddoppiati. I prezzi all'origine sono diminuiti mediamente del 13 per la maggiore parte dei prodotti, addirittura del 35-40 per cento per il mercato dei cereali; le aziende sono sempre più indebitate e stanno incontrando difficoltà crescenti in termini occupazionali; i redditi degli agricoltori sono ovunque in calo. Allora, non si può fregiare del suo titolo il Ministro di questo Governo mentre va sui trattori a manifestare contro se stesso, senza poi produrre nessuna reale misura di rilancio del comparto. Inoltre, tutto ciò avviene perdendo completamente di vista il fatto che il provvedimento su etichettatura e tracciabilità dei prodotti, approdato in Aula qui al Senato, è scomparso misteriosamente il giorno stesso della sua trattazione.

Penso che non ci si possa limitare alle solite politiche degli annunci e degli intenti come in occasione del DPEF; servono misure reali, vere, efficaci per ridare respiro ad un comparto allo stremo delle forze. citare solo alcuni degli esempi: interventi a favore degli investimenti, ammodernamento delle strutture agricole, agroalimentari, sostegno alla ricerca finalizzata, nuove fonti agroenergetiche, tutela dei territori; bisognava aiutare i nostri imprenditori agricoli per il pagamento degli interessi sui mutui di ammortamento a 15 anni, i contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole, in particolare le piccolissime aziende. Con riguardo al settore agroalimentare, il provvedimento in esame presenta un contributo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pressoché inesistente: ignora completamente la questione dell'indebitamento delle aziende agricole; non presenta misure specifiche in materia di credito d'imposta in agricoltura; agricoltura; non menziona minimamente misure per l'accesso al credito e per l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari e della pesca, né tantomeno vi è traccia di interventi finalizzati all'attivazione e all'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali necessari a governare questa difficile fase congiunturale. mi avvio alla conclusione. Non sono minimamente affrontati i problemi del sistema assicurativo in agricoltura e il rifinanziamento triennale del Fondo di solidarietà nazionale. I dati indicano che le polizze assicurative in agricoltura hanno subito una battuta d'arresto del 15 rispetto allo scorso anno, venuta a coincidere proprio con varie calamità naturali. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che ciò a cui stiamo assistendo è una pantomima che si trascina ormai da tempo lunghissimo. Abbiamo assistito a promesse e annunci, l'ultimo del quale del collega Tremonti stamattina (collega di Zaia, ovviamente) che ha sottolineato che il Fondo di solidarietà nazionale è un problema del comparto agricolo e pertanto da risolvere prioritariamente con le risorse di competenza del Dicastero agricolo. Il nostro giudizio pertanto è molto critico sul provvedimento e non potrebbe essere diversamente dopo le considerazioni che vi ho rassegnato. L'agricoltura, colleghi, è un tema che riveste un'importanza centrale nell'agenda politica del Partito Democratico. Ci piacerebbe vedere finalmente la stessa attenzione di questo Governo, ferie permettendo.

Se non fossero stati emanati i provvedimenti del Governo, non sarebbe cambiato assolutamente niente. Anzi, in alcuni casi abbiamo appesantito il lavoro di chi sta fuori dalla politica.

con tutto il rispetto per quest'Aula e per i suoi componenti ma anche con una preoccupazione seria per il momento che vive il nostro Paese, dobbiamo dire che la richiesta, che ormai era stata già annunciata da giorni, della questione di fiducia su questo provvedimento chiude i siparietti di un teatrino di avanspettacolo di periferia dove, nel gioco delle parti, c'è un comico che non fa più ridere e vecchie ballerine che cercano, senza riuscirci, di distrarre il nervosismo degli spettatori. L'Italia incomincia a stancarsi di un repertorio di barzellette vecchio, sperimentato e consumato. Lo dico, perché non si fidino, ai colleghi parlamentari del Sud che, dopo il loro giusto richiamo a non dimenticare la fragile questione meridionale, si sono visti rispondere non con i fatti di un anno di Governo ma con un semplice annuncio che sarà varato il piano Berlusconi con una nuova Cassa per il Mezzogiorno e una nuova reiterata Banca del Sud. Così come gli abruzzesi terremotati sotto le tende, che sollevavano con dignità un grido di dolore per i loro disagi non più umanamente sostenibili, si sono sentiti rispondere di non preoccuparsi, tanto lo Stato avrebbe provveduto ad offrire loro, durante i mesi più caldi, una crociera gratis per tutti, per poi vedersi fare, con l'articolo 25 di questo decreto, la richiesta vergognosa di ripresa della riscossione dei tributi e contributi dal 1° gennaio prossimo. Non riescono a distrarre la nostra attenzione neppure i vecchi balletti del ministro Tremonti che, dopo avere avviato le due operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici, ha dovuto riconoscere che l'operazione era stata fallimentare milleproroghe ha dovuto porre in liquidazione il patrimonio di SCIP 1 e SCIP 2 con il rimborso di tutte le passività accumulate per un danno ai conti pubblici di oltre un miliardo e 700 milioni. Il Ministro ieri in Commissione è venuto a dirci che non sarà modificata la tassa sull'oro della Banca d'Italia, ma anche di non preoccuparci, perché è probabile che non venga applicata: non avevamo dubbi al riguardo.

Ci vengono però imposti tempi contingentati per esaminarlo, migliorarlo e correggerlo, al punto che, come Senato della Repubblica - lo dico lo dico alla Conferenza dei Capigruppo - in proporzione abbiamo impiegato più tempo per decidere se fosse opportuno che Gheddafi entrasse o meno in quest'Aula o se la febbre suina non dovesse preoccupare gli italiani

è questa infatti la stima della Banca d'Italia di coloro che hanno lavori atipici e parasubordinati, senza diritto ad alcun tipo di protezione sociale; dei 700.000 giovani del Meridione - e questi sono dati dello SVIMEZ ‑ laureati o con altri titoli di studio che abbandonano la loro terra per trovare nuove possibilità. Questo è anche il Sud, il nostro Sud: prima emigravano le povertà ed i bisogni, oggi sono costrette ad emigrare le intelligenze e le risorse. Com'è stato detto da tanti colleghi che mi hanno preceduto, questo decreto è infarcito di errori, articoli incoerenti e norme sconclusionate; ci viene detto, però, che non è possibile correggerlo, perché più che salvacrisi, è un decreto salvaferie, o meglio, salvamaggioranza, perché l'estate servirà a guadagnare tempo per calmare le tensioni sempre più destabilizzanti all'interno del centrodestra. E poi il Governo, prima ancora che venisse approvato questo provvedimento, che doveva rispondere ad uno stato di necessità e urgenza, aveva già annunciato che ne sta preparando un altro per correggerlo. Nel nostro ordinamento costituzionale - lo dico all'amico Li Gotti, che è giurista esperto - introduciamo così una nuova formula: il decreto correttivo, detto anche il decreto-*bis*. Crediamo si confermino due questioni e si aprano due partite importanti, la prima delle quali è politica: per un Governo che gode della più ampia maggioranza numerica della storia repubblicana, sudditanza del potere legislativo a quello esecutivo diventa il manifesto politico di questo centrodestra, ed è il manifesto di un nuovo moderno regime. E ogni volta che il Governo decide di ricorrere alla questione di fiducia sembra sentire nuovamente rimbombare in quest'Aula i giudizi di fastidio e insofferenza pronunciati da Berlusconi a proposito delle Camere che, nel migliore dei casi, perdono tempo,

e in due ore di Commissione? Mentre Tremonti si diletta alle mancate stabilizzazioni dei conti pubblici, mancano a questa maggioranza una visione organica ed un progetto complessivo, perché non trova la soluzione nell'individuazione delle priorità e nella collegialità delle scelte. E tutto questo a loro non possiamo darlo noi: le liti tra Ministri non sono la febbre, ma la malattia dell'Esecutivo e la sindrome dell'uomo solo al comando non è un ripiego per il decisionismo e la tempestività delle scelte, ma la cultura ideologica di una nuova sovranità. Una seconda considerazione è sostanzialmente economica, perché, quando si manifesta - com'è avvenuto in questo decreto - una linea di politica economica ben precisa, che non tiene conto delle condizioni sociali del Paese e non fa ciò che sarebbe necessario per renderle meno sofferte, si possono seguire soltanto due possibilità. O si ha il coraggio di incidere sul bilancio pubblico, anche mettendo a rischio gli equilibri dei conti che già non vi sono, oppure si mettono a repentaglio equilibri ben più importanti, che sono quelli sociali: e ciò significa prepararsi ad affrontare nel prossimo autunno un serissimo problema di tenuta sociale.

e le risorse che vengono presentate come aggiuntive, come quelle per gli ammortizzatori sociali, non sono affatto adeguate a tassi di disoccupazione a due cifre. Questo significherà in sostanza che il Governo dovrà intervenire di nuovo in corso d'opera, in una manovra finanziaria permanente e continua - siamo ormai all'ottavo decreto-legge anticrisi - per ridurre l'entità delle erogazioni oppure per migliorare le dotazioni dei vari fondi, agendo di nuovo e tardivamente e rendendo ancor più distorsivi gli effetti della spesa pubblica.

Ce lo spiega la stessa relazione del Servizio bilancio del Senato facendoci alcuni esempi: un miglioramento dell'indebitamento netto è connesso alla regolarizzazione delle badanti - pensate, guadagniamo con le badanti! e viene utilizzato per incrementare la spendibilità nell'adozione delle delibere CIPE di assegnazione delle risorse FAS attivate a favore dell'Abruzzo. Analogamente, anche l'Abruzzo fa la sua parte. Dopo la sospensione dei versamenti fiscali a favore dell'Abruzzo, la richiesta di recupero immediato dei tributi a partire da gennaio viene registrata tra le maggiori entrate. Per il 2009 il CNEL prevede Per il 2009 il CNEL prevede un bilancio finale rovinoso sul piano dell'occupazione, calcolata in forze di lavoro - per capirci, persone in carne ed ossa - cacciate dalla produzione, in una forchetta che va dalle 350.000 alle 540.000 unità. Poco spazio, ma non certo solo di ordine temporale ma anche di volontà politica - mi permetto di ricordarlo a quei colleghi con l'orologio in mano in Commissione in mano in Commissione - hanno trovato le nostre proposte di rafforzamento degli ammortizzatori sociali, di allargamento della regolarizzazione dei lavoratori stranieri, di una fiscalità di vantaggio per il Sud, mentre gli esponenti di questa maggioranza hanno preferito ancora una volta concentrarsi sull'ennesimo condono che premia chi evade, chi viola la legge, chi inganna i cittadini onesti che pagano le tasse, sino ad arrivare alla vergogna delle vergogne che prevede la restituzione al fisco delle tasse a partire dal prossimo anno per i terremotati sotto le tende e senza casa in Abruzzo. Questa è la situazione. Voglio ora entrare nel merito di alcuni punti. L'articolo 1 doveva essere l'articolo che allargava gli ammortizzatori sociali ad una platea più ampia di lavoratori, mentre sarà invece l'articolo che allargherà le ingiustizie e le disuguaglianze, momento che la misura più importante, che prevede di far restare i lavoratori a frequentare corsi di formazione forniti dalla loro azienda, non può certo migliorare le opportunità di impiego di quei lavoratori che sono occupati in quelle tante imprese che non hanno un futuro oltre la crisi. Nessun intervento per quei lavoratori che svolgono lavori flessibili e che non godono di un sistema di *welfare* degno di questo nome. Rimarrà quindi un misero *spot*

mettendo paletti talmente assurdi che alla fine solo 1.800 lavoratori ne hanno potuto usufruire rispetto ai circa 400.000 precari che vedranno scadere il loro contratto di collaborazione entro l'anno. Ma non c'è solo questo. Alla copertura degli oneri derivati dall'articolo 1 si provvede con la riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione, alimentato a sua volta con le risorse del Fondo per la aree sottoutilizzate. Questo fondo, lo ripetiamo ancora una volta, non è costituito da stanziamenti aggiuntivi ma da risorse sottratte al Sud. Un altro dei punti presentati come più significativi di questo decreto legge, l'articolo 5 sulla detassazione degli utili reinvestiti, non è altro che un provvedimento che produrrà, per come è fatto il nostro Paese, un effetto di allargamento delle differenze, perché, dei 2 miliardi stanziati per questo articolo, di fatto è come prevedere che oltre 1 miliardo e 800 milioni andranno alle zone forti del Paese, avvantaggiando le grandi industrie e penalizzando le imprese piccole e medie che compongono il fragile tessuto produttivo del nostro Mezzogiorno. Siamo agli antipodi dei più elementari criteri di incentivazione allo sviluppo. Lo sgravio non viene concesso all'imprenditore che decide di puntare sulle aree depresse o sulla ripresa della sua azienda, ma premia chi ha già i risultati migliori. Cosa dire poi del *rebus* del FAS, il sistema di scatole cinesi ideato dalla genialità del ministro Tremonti? Non ci hanno convinto i conticini fatti dal sottosegretario Giorgetti in Commissione e noi dell'Italia dei Valori aspettiamo un'informativa del Governo sul quadro delle risorse di competenza ancora disponibili, sul Fondo nazionale e sulle risorse di casa effettivamente disponibili da qui al 2013. Cosa dire, ancora, sulla palese incostituzionalità dell'articolo 17? Infatti, in un decreto economico, caro collega Li Gotti, finiscono norme sulla Corte dei conti che non hanno alcuna compatibilità con il tema generale e non rivestono carattere di necessità e di urgenza. Non mi soffermo poi sulla foglia di fico dello scudo fiscale dell'articolo 13-*bis*, perché lo stesso Governo ha piena coscienza della negatività di questo intervento, al punto che si è voluto in tutti i modi mascherare il provvedimento sotto mentite finalità benefiche, collegandolo, da un lato, alla repressione dell'utilizzo dei paradisi fiscali

tre correzioni: sulla Corte dei conti, sulle competenze del Ministero dell'ambiente e ritocchi allo scudo fiscale. Continua quindi la manovra infinita che, per il momento, ha forse dato qualche

della crisi stessa nei termini che conosciamo. Si emanano provvedimenti; i dati relativi all'andamento dell'economia, dell'occupazione, del PIL, dei conti pubblici si aggravano: si emana un altro provvedimento; quei dati si aggravano ancora: si emana un altro provvedimento, e così via. Un avvitamento sempre più evidente che scopre l'inefficacia della politica complessiva del Governo nel contrastare la più grave recessione dal dopoguerra ad oggi. Ciò che rileva, sotto questo profilo, non è tanto la valutazione dei singoli provvedimenti e delle singole misure che pure possono essere, almeno per una parte di loro, condivise: se si riconosce il credito d'imposta piuttosto che misure implementative degli ammortizzatori sociali, come non condividerle? Ciò che rileva e che abbiamo cercato di dire in questi giorni, e che voglio ora ribadire, è che gli effetti macroeconomici del complesso delle misure adottate dal Governo, e quindi anche di questo decreto, sono molto limitati, sono ben poca cosa rispetto all'entità, al volume dei problemi che abbiamo di fronte.

6 per cento. L'anno prossimo, l'incidenza delle misure anticrisi sul prodotto interno lordo si fermerà allo 0,44 per cento. Questi sono i fatti, i dati forniti dal Governo, ripeto, che ci dicono appunto che il volume

quelli che si devono ancora manifestare, sono ulteriormente devastanti, non solo sul PIL, ma anche - come abbiamo visto - sulla disoccupazione, soprattutto,

può tentare di occultare. Ma i dati, i fatti, le sofferenze, i problemi, le incertezze, le insicurezze, le debolezze della nostra economia e della nostra società sono sotto gli occhi di tutti. L'atteggiamento del Governo è: «La crisi passerà», ma gli effetti - diciamo noi - sono ancora destinati a manifestarsi in senso negativo sul piano sociale, sociale, occupazionale e sui conti pubblici. Nel merito delle singole misure è stato detto molto, in questo dibattito, e io non voglio aggiungere nulla

Mi preme soltanto tornare su un tema, che è stato molto presente nella discussione e che necessita di qualche precisazione e affermazione più chiara e più precisa, quello delle tasse dei terremotati. si è tanto discusso nell'altro ramo del Parlamento e poco in questo ramo del Parlamento, perché ‑ come è noto ‑ siamo stati costretti ad una discussione angusta in Commissione e poi a questo dibattito in Aula, che si sta svolgendo nei modi che vediamo, senza sufficiente attenzione. Anzi, ringrazio i pochi colleghi presenti, perché stanno qui ad ascoltare e a seguire la discussione su un provvedimento così importante.

non pagati quest'anno. Il decreto stabilisce la copertura delle minori entrate, nell'anno in corso, per 513 milioni di euro e l'utilizzo delle maggiori entrate previste per il 2010 e il 2011 per finalità legate alla copertura di questo decreto. Tradotto: i 513 milioni che gli abruzzesi riverseranno o dovranno riversare l'anno prossimo e quello successivo nelle casse dello Stato serviranno a pagare le misure anticrisi del Nord e del Sud, ma prevalentemente del Nord, dato che gran parte del tiraggio - come si dice - della

Vi sono state numerose proteste da parte della popolazione e delle istituzioni locali e una chiara presa di coscienza da parte di tutte le forze politiche, anche di maggioranza. Piuttosto che cambiare il decreto in Aula alla Camera o qui in Senato, il Governo si è affidato ad una promessa verbale. Non è la prima volta che questo accade, ma qui sta accadendo in un modo che è senza precedenti, cioè il Ministro dell'economia, il sottosegretario Bertolaso e poi il sottosegretario Giorgetti in Commissione ieri sera, hanno detto che questa legge, che oggi stiamo approvando, sarà cambiata con un'ordinanza, cosa che non è mai accaduta prima e che pone enormi problemi. Tralascio la mostruosità giuridica sottesa ad una scelta di questo tipo, cioè: nel giorno nel quale si approva una legge dello Stato, il Governo dice ufficialmente che la modificherà o l'abrogherà con una ordinanza. Tralascio questo aspetto e voglio invece sottolineare i problemi finanziari: se le nuove entrate previste per effetto di questa odiosa misura sono portate, come ho detto, a copertura delle misure recate nel decreto, quando si tratterà di emanare un'ordinanza, che come è noto non è una legge, come si coprirà quella ordinanza? Cioè, come si garantirà la copertura finanziaria dell'auspicato promesso nuovo differimento delle imposte? Questa è la domanda che abbiamo rivolto. A questa domanda il Governo non ha risposto, perché non può rispondere perché è vera una sola cosa, cioè che, se non cambierà la legge (e per questo ci auguriamo che le modifiche preannunciate contengano questa misura, anche se ho molti dubbi che ciò avvenga, perché bisognerà appunto trovare in pochi giorni

una doppia rapina a danno degli abruzzesi: prima si destinano le imposte, precocemente richieste loro, alle finalità del decreto; dopo, se sarà l'ordinanza di protezione civile a provvedere in materia, si chiederà loro di sopportare una decurtazione dei fondi stanziati per il terremoto. Mi dispiace che oggi il presidente Quagliariello si sia cimentato in un'operazione, signor Presidente, di commento di forti preoccupazioni che io ed altri senatori, tra cui il senatore esposto anche sull'elemento che è emerso ieri sera in Commissione, cioè che i famosi 4 miliardi per la ricostruzione provenienti dal FAS, in realtà, non sono subito disponibili. Lo ha detto il Governo:

sottolineatura del fatto che per un anno e mezzo avremo fondi di scarsissima entità, il presidente Quagliariello si è cimentato in una reazione scomposta e offensiva (e me ne dispiaccio fortemente), apostrofando chi parla e il senatore Lusi come protagonisti di un'accozzaglia di falsità, come persone intente a lucrare briciole di visibilità sulla pelle dei terremotati, che negano l'evidenza.

La verità è che in Abruzzo si sta facendo molta propaganda, molta pubblicità, molta ostentazione e si sta provvedendo con le famose casette, mentre di ricostruzione si parlerà quando se ne quando se ne parlerà, cioè, nella migliore delle ipotesi, dal 2011 in poi. Questa è la verità. Rispondete a queste obiezioni, a queste domande, a queste preoccupazioni nell'interesse di quei cittadini, dopodiché confronteremo le reciproche posizioni. Non rendetevi protagonisti di falsità, menzogne e insulti,

Signor Presidente, signor Vice ministro, onorevoli colleghi,

anche alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi dell'opposizione, che mi sono convinto ancora di più della bontà del provvedimento che, se non sarà certamente rispetto agli obiettivi che ci siamo dati, appartiene a quella cornice di interventi che servono e che mano a mano, come un grande *puzzle*, stiamo ponendo in essere per far sì

ma alcune considerazioni sul terremoto, caro collega Legnini, non credo possono essere usate nei confronti del Governo Berlusconi. Io, che vivo in Campania e che ho vissuto il terremoto del 1980, posso assicurare il collega Legnini che ancora non abbiamo completato la ricostruzione, probabilmente anche per gravi, gravissime carenze della classe politica campana, specialmente di sinistra.

Credo che sia ingiusto e ingeneroso rivolgersi in questo modo al Governo sul problema dell'Abruzzo. Credo che sia una delle punte di diamante del Governo e del nostro presidente Berlusconi, al di là dell'appartenenza a questa parte politica. Al riguardo, dunque, vorrei invitare i colleghi dell'opposizione, soprattutto gli abruzzesi, ad essere più sereni nell'esaminare quello che sta facendo il Governo, a suggerire eventuali modifiche ed interventi di sostegno ulteriori a questa azione; ma certamente

vorrei soffermare l'attenzione: a situazioni negative non si sarebbe potuto rispondere con ulteriori aggravi di pressione fiscale sulle famiglie e nuovi incrementi di spesa pubblica improduttiva; e non lo abbiamo fatto. le risorse, per una parte mediante mirati incrementi delle entrate, per nulla a carico delle famiglie, e, per altra parte, con riduzione degli degli sprechi, in maniera particolare riducendo la spesa farmaceutica. La scelta del Governo, confermata con il decreto-legge n. 78 al nostro esame, è stata dunque sin dall'inizio in controtendenza a tante scelte di decenni passati; è stata tesa a salvaguardare quantomeno gli andamenti a legislazione vigente, a non peggiorare, cioè, i saldi di finanza pubblica più di quanto faccia già la fase recessiva. Fortunatamente la fase negativa del ciclo volge al termine: lo stiamo ripetendo da più tempo creando anche entusiasmo; qualcuno, della sinistra soprattutto, ci ha tacciato di essere degli illusionisti e degli illusi sulla ripresa dell'economia: invece - lo stiamo vedendo - cominciamo vedendo - cominciamo ad uscire dalla curva o dal tunnel. E lo stesso Obama, qualche ora fa, ha dichiarato che anche gli Stati Uniti si stanno avviando in questa direzione. Certo, purtroppo per il Sud, Sud, per noi altri, permangono elementi di preoccupazione. Vi sono una serie di fattori esogeni che ci affliggono ed avviliscono. Una politica antica non è riuscita a creare le condizioni

la Cassa per il Mezzogiorno, da una felice intuizione di Pasquale Saraceno, che non era certo meridionale ma che aveva voluto vedere in quello strumento la capacità di accompagnare nel dopoguerra il nostro Paese. Ebbene, oggi,

è riuscito a creare le condizioni affinché per davvero fosse fugata l'idea di un Nord contro il Sud e di un Sud piagnone. Ci avviamo per davvero, con l'accordo fatto già con la Regione Sicilia

la Regione Campania, devo comunicarlo, è riuscita a spendere appena il 17 per cento dei fondi 2001-2006, quindi, nemmeno questo riescono più a fare. Finora il presidente Bassolino, con la giunta di sinistra, ha dilapidato risorse incredibili, senza creare le precondizioni dello sviluppo, senza cioè dotare il nostro territorio di una infrastrutturazione

modernizzare i sistemi informativi per una maggiore efficienza e una trasparenza degli uffici pubblici; ha invece rivolto la spesa verso determinati obiettivi tipici della sinistra ed anche, per la verità, nel passato, della vecchia Democrazia Cristiana (che aveva creato soltanto un apparato di sostegno per governare i processi e gli enti e non creare le condizioni dello sviluppo). Occorre anche sostenere fortissimamente il turismo, nel Mezzogiorno d'Italia.

affinché il nostro Paese possa riprendersi, svilupparsi e camminare nel migliore dei modi. Noi siamo convinti che il Governo del presidente Berlusconi questa maggioranza siano, non soltanto nelle condizioni, ma nella ferma e determinata convinzione che con questo faremo il bene del Paese. Finora lo abbiamo fatto e lo continueremo a fare.

*(IdV)*. Signor Presidente, come avevo preannunciato all'inizio della seduta, oggi il Consiglio dei ministri ha deliberato di riconsiderare la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Fondi, sulla base di una nuova relazione che lo stesso ministro Maroni dovrà sottoporre al Consiglio dei ministri, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Questo è l'ennesimo schiaffo alla legalità e alla democrazia che poteva dare questo Governo. Di fatto, con questa decisione del Consiglio dei ministri siamo tornati indietro, perché il ministro Maroni sarà costretto a scrivere una nuova relazione da sottoporre al Consiglio dei ministri al fine di poter finalmente sciogliere il Consiglio comunale. Oltretutto, la motivazione è assolutamente falsa perché, caro Presidente, la nuova legge n. 94 del 2009, addirittura citata dal Consiglio dei ministri, entrerà in vigore

non è vero che non possono sciogliere il Consiglio comunale di Fondi: in realtà non lo vogliono sciogliere perché qualcuno che siede lì, al Consiglio dei ministri, su quel tavolo, è colluso con la criminalità.

dovremmo concludere, signor Presidente? Che fra i 24 Ministri (includendo anche il sottosegretario Letta) che siedono in Consiglio, oggi ci sono state delle belle novità: o è stato creato un venticinquesimo Ministero per la tutela della criminalità organizzata oppure a qualcuno dei Ministri attuali è stata data la delega alla protezione dei mafiosi. Il problema essenziale è che davvero qualche nome eccellente protegge i mafiosi. E io voglio sapere chi è, perché gli atti sono secretati. Lo chiedo al Presidente lo chiedo al collega Fazzone, più volte nominato nelle cronache, lo chiedo a Tajani, lo chiedo all'UDC, perché il loro tacere, il loro difendere genera dubbi e io spero sempre

qualche nome eccellente protegge questi mafiosi. Allora - e con questa amara conclusione concludo - ho denunciato tanto il silenzio colluso del Governo, ma forse quel silenzio mafioso era, seppur grave, migliore delle bugie di questo Governo, che sono offensive per i cittadini, per il prefetto Frattasi e per il ministro Maroni, che ora è obbligato a riscrivere l'intera vicenda dello scioglimento solo per prendere tempo e per garantire alla criminalità organizzata di festeggiare ancora una volta, perché protetta da qualcuno che siede in quel Consiglio dei ministri. Senatore Pedica, naturalmente la Presidenza prende atto del suo intervento. Lei ha a disposizione anche strumenti di sindacato ispettivo, se vorrà utilizzarli, per avere risposte specifiche.